la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità alcune modifiche al calendario corrente, stabilendo anzitutto di trasferire presso le Commissioni riunite esteri e difesa - nella data che le Commissioni medesime concorderanno con il Governo - le comunicazioni previste in Aula per oggi pomeriggio, al fine di consentire una più ampia trattazione delle tematiche connesse alla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Per il resto rimane confermato il calendario, salvo gli orari della seduta antimeridiana di giovedì 19 aprile (dalle ore 9 alle ore 11,30) e la ripresa dei lavori, nella settimana successiva alla prossima, a partire dalle ore 16 di mercoledì 2 maggio. È stato ribadito che la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha dato mandato al Presidente di valutare, in relazione all'andamento dei lavori e al *quorum* richiesto, la data di inserimento delle votazioni per il diniego di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Marzano e degli altri coimputati.

mi ero premurato di chiedere ad alcuni Capigruppo di tenere in debito conto il fatto che per la giornata di domani pomeriggio è prevista una manifestazione della Costituente per il partito democratico, onde tentare, eventualmente,

nella seduta pomeridiana di domani non abbiano inizio prima delle ore 18,30, in considerazione del fatto che la nostra manifestazione avrà inizio domani, alle ore 16, in piazza Montecitorio. È evidente, signor Presidente, che la nostra richiesta confida anche sulla cortesia istituzionale e sulla disponibilità di tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

per il futuro, ma abbiamo valutato lo svolgimento dei congressi e abbiamo fissato i tempi a voi comunicati oggi pomeriggio. Resta il fatto che iniziative diverse

È questo un aspetto molto significativo e importante, nel senso che nel Senato e tra i Gruppi parlamentari del Senato c'è una consapevolezza che il bene prodotto agricolo può essere difeso se c'è una convergenza

L'agricoltura italiana si difende, rispetto alla competizione all'interno della Comunità Europea che non sempre è propensa ad accogliere e a rispondere

unitari ad un consapevole voto sulla mozione presentata, il Governo chiede che la votazione avvenga per parti separate.

il Governo prende atto che, da parte dei Gruppi parlamentari, vi è una posizione unitaria e positiva per affrontare e risolvere i grandi problemi dell'agricoltura.

Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per esprimere il nostro voto sulle mozioni n. 51, 68 (testo

già anticipato nel corso degli approfonditi lavori della Commissione agricoltura, hanno dimostrato una sostanziale unitarietà di intenti tra maggioranza e opposizione per ciò che riguarda le problematiche e gli impegni che il Governo dovrà assumere nel settore agroalimentare, in particolare sull'industria conserviera del pomodoro e dei prodotti ortofrutticoli. Voglio, quindi, porre l'accento, essendo già intervenuto sul merito delle mozioni in sede di discussione generale, sulla positività dei comuni intendimenti su alcuni fondamentali aspetti della nostra agricoltura, di politica agricola comunitaria ed internazionale; aspetti fondamentali dal punto di vista sociale, economico ed ambientale del nostro Paese ed in particolare per lo sviluppo del Mezzogiorno. È bene, infatti, che vi sia un sostegno comune di queste mozioni orientate a favorire processi di concorrenza leale e di trasparenza e indirizzate, per mezzo della predisposizione di sistemi a garanzia dell'alta qualità dei prodotti e del rispetto delle norme igienico sanitarie,

che stiamo parlando di un settore che non è in via di dismissione, come qualcuno pensa, ma di un settore ancora fondamentale per l'economia del nostro Paese. Il settore agroalimentare è il secondo comparto in Italia e

se non ha dietro di sé un forte settore agricolo. Questo lo dobbiamo sapere. Quindi, è una battaglia che deve vedere coinvolto tutto il Paese. Devo dare atto al ministro De Castro che recentemente, anche nell'incontro con il suo collega spagnolo,

Credo che da questo punto di vista abbiamo le carte in regola, perché l'Europa dice, con chiarezza, che non si può indicare l'etichettatura, a meno che non vi sia un errore in cui verrebbe indotto il consumatore. Nel nostro caso, credo che di errori ve ne siano moltissimi e che su questi si si alimenti un vasto mercato della contraffazione. Sapete perfettamente che nelle esportazioni (soprattutto negli Stati Uniti) sono più i prodotti contraffatti come *made in Italy*

Ferrero, che ha pensato di prevedere etichette sugli alcolici, per ricordargli che il vino è un nostro settore di punta per l'esportazione e che non ha nulla a che fare con altri danni le altre mozioni, è importante che il Senato si sia espresso e abbia discusso alla vigilia di una riforma così importante come quella dell'OCM ortofrutta, un settore in cui credo l'Italia occupi buone posizioni. Vorrei ricordare che per il pomodoro siamo i secondi produttori mondiali e che sull'ortofrutta eravamo, fino a poco tempo fa, forse i primi. In questo senso bisogna andare avanti con serietà non assumendo atteggiamenti che possono essere preclusivi degli interessi del comparto.

perché - ripeto - su alcuni settori dobbiamo essere cauti. Al contrario del senatore Scarpa Bonazza Buora, anch'io ero molto perplessa - devo dire che ho mantenuto alcune mie perplessità - sulla scelta del disaccoppiamento totale, perché nel campo dei cereali ci è costato e credo ci costerà ancora.

il futuro industriale del Paese in questo settore: abbiamo un presente industriale nella trasformazione, soprattutto del pomodoro, e siamo - mi auguro ancora a lungo - il secondo Paese produttore del

un rapporto di correttezza in tutta Europa e quindi abbiamo chiesto al Governo, nella trattativa per l'ortofrutta a livello europeo, di dare quello che è uno dei nostri contributi: un rapporto trasparente con il consumatore. Noi vogliamo che sia scritto sull'etichetta da dove proviene il pomodoro che gira per l'Europa: se è pomodoro cinese, che sia scritto che è cinese; se è pomodoro italiano, che sia scritto che è italiano. È una È una piccola rivoluzione, che costa poco, ma che consentirà di mantenere la nostra industria di trasformazione. In secondo luogo, abbiamo chiesto dei compartimenti stagni, nel senso cioè che nella ripartizione dei fondi europei

di identificare risorse certe, magari anche aggiuntive, da parte del Governo, per poter mantenere la nostra industria,

non ha raggiunto un buon livello di trasparenza produttiva e che deve camminare con le sue gambe mantenendo un migliore rapporto con la produzione.

favore della mozione del collega Scarpa Bonazza Buora, che parla di disaccoppiamento totale. Il Governo ha identificato la forma del crediamo sia un compromesso accettabile, tenendo presente che c'è una parte del Paese che è in grado di reggere il disaccoppiamento totale ed un'altra che ancora oggi non potrebbe reggerlo. È una soluzione di compromesso intelligente

Tutte le mozioni, infatti, sia pure con sensibilità e sfumature diverse, pongono l'accento su due problemi fondamentali dell'agricoltura italiana: quello del mantenimento dei livelli di qualità (quindi, la tutela della qualità del prodotto italiano) e quello conseguente alla riforma dell'OCM ortofrutta e quindi il disaccoppiamento. In particolare, il problema dell'etichettatura, trattato nella mozione De Petris anche a proposito dell'olio d'oliva, è ripreso dalla mozione Polledri per quanto attiene la provenienza del pomodoro trasformato. Da sempre il pomodoro è un *testimonial* nel mondo del *made in Italy* ed Alleanza Nazionale è particolarmente preoccupata che, in occasione, appunto, dell'applicazione del disaccoppiamento, possano unirsi le sorti degli agricoltori e quelle degli industriali, verificandosi da una parte un calo di produzione e, quindi, la diminuzione degli occupati in agricoltura, dall'altra la riduzione degli impianti di trasformazione che già nell'ultimo quinquennio sono diminuiti del 20 per cento: da 200 sono diventati 180. Per quello che attiene al disaccoppiamento, le soluzioni lievemente diverse proposte dalla mozione a prima firma presentata dal senatore Scarpa Bonazza Buora dimostrano quali diverse problematiche possiamo incontrare in giro per l'Italia relazione all'eventualità dell'immediata applicazione del disaccoppiamento. Alleanza Nazionale ritiene che, o un breve ritardo

*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto mi sia consentito rivolgere un ringraziamento affettuoso e sincero al collega Polledri che ha voluto ricordare la mia modesta esperienza di Governo. Passando al punto che è stato ampiamente trattato durante la seduta di giovedì scorso, mi piace ricordare che abbiamo svolto un dibattito sicuramente molto approfondito, sereno e allo stesso tempo particolarmente tecnico questo ci ha permesso di consolidare le nostre opinioni, confrontarle e anche - se possibile - perfezionarle, in uno spirito assolutamente unitario e positivo, atto a conferire al ministro De Castro un viatico importante, per il tramite di questo ramo del Parlamento, che lo possa rinsaldare in funzione della difficile trattativa che si terrà, di qui a qualche mese, in sede comunitaria per la riforma dell'OCM vitivinicolo

i parlamentari degli altri Paesi con grandi agricolture come la nostra: fare squadra e «quadrato», senza nasconderci le diversità che indubbiamente esistono, ma cercando di perseguire un'attività negoziale che si rivelerà estremamente complessa.

Chi mi conosce e segue il dibattito di politica agricola nazionale sa che la mia posizione e quella di Forza Italia è sempre stata, negli anni precedenti alla riforma di metà periodo della politica agricola comunitaria,

in modo anticipato pressoché dalla totalità dell'opinione politica agricola nazionale e comunitaria, in particolare dall'allora commissario europeo all'agricoltura Franz Fischler nel 2002-2003. Fischler nel 2002-2003. Forse sarebbe stato opportuno attendere prima la conclusione dei negoziati WTO e, secondariamente, andare a fare una derivata e quindi costruire ed applicare una politica agricola comunitaria che potesse reggere nel tempo. Noi, invece, abbiamo fatto esattamente il contrario:

Manteniamo la nostra impostazione favorevole al disaccoppiamento totale, sapendo che oltretutto sulla nostra posizione, si ritrova gran parte degli agricoltori italiani, rappresentati dalle grandi organizzazioni storiche dell'agricoltura italiana, innanzitutto Coldiretti e Confagricoltura. Quindi, gran parte delle organizzazioni agricole del Paese in questo momento stanno guardando con attenzione alla posizione di Forza Italia e questo ci conferma nella convinzione di aver fatto bene a mantenere questa posizione. Non mi dilungo sugli altri aspetti della nostra mozione, perché ampiamente trattati negli interventi di giovedì scorso. Annuncio che certamente sosterremo con la massima convinzione, senatrice De Petris, la sua sua mozione riguardante l'etichettatura obbligatoria. È una posizione tradizionale, anche nostra, ma credo che sia una posizione totalitaria del Senato, dell'intero Parlamento e delle forze politiche italiane. È certamente un'impostazione totalitaria degli agricoltori italiani, che hanno bisogno di vedere difesi i propri prodotti senza misure protezionistiche, ma con misure che diano spazio alla valorizzazione della qualità del *made in Italy*, del prodotto in campagna dall'impresa agricola del nostro Paese. Questa è una battaglia comune dell'Italia, una battaglia forte che abbiamo sostenuto anche ad Hong Kong quando ci siamo recati per le trattative, purtroppo conclusesi con un insuccesso, un anno e mezzo fa. Ricordo che allora l'Italia era molto isolata a livello comunitario. Ricordo i Consigli europei durante i quali

ad uniformarci a questo tipo di impostazione: quindi, certamente disaccoppiamento totale, ma con qualche accorgimento. Qualcuno dice di prorogarlo nel tempo; io dico semmai di mettere in atto ogni strumento utile a fare in modo che la filiera non sia

che in questa occasione, nel momento di una riforma estremamente difficile dell'Organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, che rappresenta il 25 per cento dell'agricoltura italiana circa, abbiamo fatto un lavoro eccellente di collaborazione, franco, leale,

finestra") *(Ulivo)*. Dv Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo sia stato opportuno e tempestivo portare all'attenzione di quest'Aula le preoccupazioni che riguardano un settore importante come quello dell'ortofrutta; preoccupazioni che giungono in particolare dal settore del pomodoro da industria e dal settore agrumicolo. Le cifre che indicano il ruolo economico della produzione ortofrutticola sono già state indicate nei testi delle mozioni e bastano ad illustrare l'importanza del comparto per l'intera economia italiana. Un settore, quello dell'ortofrutta, che rappresenta al tempo stesso: eccellenti realtà industriali di trasformazione; produzioni fortemente radicate nei territori; identità territoriali che non si misurano solo in fatturati, ma sono realtà che hanno modellato territori e paesaggi, stratificato tradizioni produttive di comunità nelle nostre Regioni del Sud e del Nord, che rappresentano valori non solo economici ma sociali e culturali (realtà che oggi sono attraversate da forti mutamenti, da esigenze di cambiamento del tutto inedite). Un settore che indica una dimensione importante in quantità di lavoro, in numero di addetti, significativo nella produzione e nella trasformazione. Alla luce di questo quadro, è particolarmente importante oggi questo dibattito, queste prese di posizione, perché significa inserirsi autorevolmente in un confronto in tempo reale con l'Europa, che si sta accingendo a varare a breve una delle importanti riforme (assieme alla riforma del settore vitivinicolo): la revisione dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta; una riforma nella quale il nostro Paese, nel cuore del Mediterraneo, ricco di eccellenze di produzioni ortofrutticole, può e deve portare (in alleanza con altri Paesi mediterranei), scelte innovative capaci di incidere sugli indirizzi europei per una valorizzazione delle produzioni, specificità nazionali dei territori di produzione. Il settore ortofrutticolo, come peraltro altre colture mediterranee, è già stato in passato penalizzato dalle regole comunitarie, della politica dei prezzi e dei mercati rispetto a produzioni continentali. Ora la nostra posizione non è di contrapposizione all'architettura complessiva della riforma: com'è stato detto nel dibattito, ne condividiamo obiettivi generali e finalità. È condivisibile che si possa allargare al settore ortofrutta la strategia europea imboccata negli altri settori: politiche tese a ricondurre tutte le organizzazioni di mercato nel regime di pagamento unico aziendale ovvero a potenziare la capacità competitiva, l'orientamento al mercato, a rendere le produzioni sostenibili sia nel mercato interno che sui mercati esteri. Non c'è dubbio: se si vuole dare prospettiva imprenditoriale, occorre passare sempre più dalla logica del sostegno alla produzione (che purtroppo spesso ha significato produrre per il sostegno)

del sistema dell'aggregazione per l'immissione sui mercati. Quindi, non c'è dubbio che un cambiamento di impostazione sia indispensabile. Tuttavia, come emerso da più interventi, non si condivide (vi è una forte preoccupazione la proposta di un passaggio immediato al cosiddetto disaccoppiamento totale, che porterebbe alla disarticolazione di interi settori e filiere, come quella del pomodoro, con conseguenze fortemente negative per l'occupazione e la stessa solidità delle filiere. Riteniamo (anche in coerenza con le riforme europee fin qui approvate) sia indispensabile un adeguato periodo di transizione e di adattamento non traumatico, che tuteli i produttori storici di ortofrutta e li accompagni nella nuova fase. Devono infatti essere guardati con altrettanta attenzione i segnali che provengono da rilevazioni statistiche ed economiche per cui il disaccoppiamento totale ha provocato l'abbandono di territori, con conseguente effetto di degrado sociale e ambientale. In quest'ottica evidenziamo con preoccupazione la situazione che si è determinata nella coltura degli agrumi, in aree spesso fragili sia dal punto di vista ambientale che economico. Il nuovo sistema, con un approccio immediato del disaccoppiamento, avrebbe come conseguenza di far scomparire diverse industrie, che, per dimensioni e per scarsa forza di strutture aziendali, richiedono percorsi e tempi adeguati per le riconversioni, per quelle innovazioni che riteniamo assolutamente indispensabili. Pertanto, vogliamo invitare l'Unione Europea ad una riflessione approfondita sulle conseguenze delle proposte avanzate; ad una coerenza reale - come è stato detto - tra obiettivi enunciati dalla Commissione e risultati a seguito delle misure previste, la coerenza finanziaria soprattutto. Solleviamo perplessità quando si introducono nuovi importanti misure nei programmi operativi, che condividiamo, misure innovative ma che, combinate con la permanenza di vincoli percentuali alla partecipazione di programmi operativi, portano a un'obiettiva diminuzione di risorse disponibili per gli investimenti e l'occupazione nel settore. Di fatto, questo non rispetta il principio di invarianza di bilancio enunciato; di fatto si penalizza un settore che, al contrario, deve trovare risorse, misure, criteri per raggiungere le finalità enunciate: un'aggregazione dell'offerta per gestire al meglio le sfide del mercato e per ridurre la frammentazione del sistema agroalimentare; stabilizzare il reddito dei produttori e ridurre quelle incertezze e fluttuazioni che spesso sono causa di ostacolo all'ingresso di giovani imprenditori nel settore; tutelare l'ambiente e l'ecosistema con adeguati sistemi di produzione; promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli. Riteniamo giusto e auspicabile che misure e azioni prevedano un potenziamento delle organizzazioni dei produttori come strumento di concentrazione dell'offerta e, ancora, un coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori nella gestione delle crisi di mercato, con destinazioni di *budget* e risorse non all'interno delle risorse esistenti ma con risorse ulteriori. C'è poi una domanda di equo rigore che arriva dal nostro sistema produttivo, sistema che proprio sulla qualità, sulle garanzie di provenienza e di corretti procedimenti di trasformazione, sulla sicurezza alimentare e l'informazione trasparente al consumatore vuole giocare il proprio futuro in Europa e nel mondo, come carattere distintivo, come carta d'identità del *made in Italy* agroalimentare. Questo rigore nei controlli e negli accreditamenti dev'essere garantito e dev'essere per tutti. La sfida della competitività si può proporre, si può affrontare se è certo che si basa su regole comuni. Devono essere considerati parametri fondamentali nelle norme di commercializzazione la garanzia dei consumatori, la garanzia rispetto alla provenienza del prodotto, la salubrità e le norme igieniche. È per questo che l'Italia dev'essere convintamente in testa a quella battaglia che vuole introdurre nelle norme che regolano gli scambi internazionali la tracciabilità come misura di base per la gestione del rischio sanitario, come etica del commercio e del consumo, come diritto fondamentale alla conoscenza, ad una consapevolezza sempre crescente. Per questo condividiamo i contenuti della mozione che impegna il Governo a sostenere e a riconfermare in sede comunitaria la validità della legge n. 204 del 2004, convinti che non siamo nel campo della concorrenza sleale o di ostacoli alla libera concorrenza, ma nell'ambito del diritto all'informazione e alla trasparenza. Siamo di fronte a un provvedimento volto ad assicurare un elevato livello di protezione rispetto a tutti i cittadini dell'Unione contro forme di concorrenza chiaramente sleali. È emblematico l'esempio dell'olio d'oliva di origine vergine ed extravergine, un prodotto sul quale luogo di coltivazione, luogo di raccolta, pratiche tecniche di estrazione e luogo di estrazione incidono significativamente sul risultato finale, sulla qualità, sulle caratteristiche organolettiche. Questo ci dice quanto sia importante l'informazione completa, puntuale, verso chi deve acquistare e consumare, quanto essa sia importante per rafforzare il controllo e contrastare con forza i troppi casi di frode e contraffazione nel settore ortofrutticolo e nel settore degli oli d'oliva in particolare. Chiediamo quindi al nostro Governo di portare convintamente in Europa questa che vorremmo chiamare filosofia forte di posizioni politiche unanimi, del sostegno di associazioni di cittadini, di tanti consumatori, di chi non vuole rassegnarsi e tornare indietro a considerare il settore agroalimentare unicamente una strategia produttiva e da standardizzare, ma al contrario vuole non solo riconfermare la grande opportunità che il nostro Paese ha delle grandi differenze specifiche, ma portare in Europa - anche nel nord Europa - l'idea che sempre più, in un mondo che si sta velocemente omologando, distintività, identità territoriali, consapevolezza alta dei consumatori, potranno indicare nuove sfide per l'intera Europa, potranno essere fattori decisivi per livelli innovativi di competizione. Sarà il modo per governare la globalizzazione senza rimanerne travolti e annullati. Per questo motivo,

della ex Manifattura tabacchi di Rovereto che, dopo la dismissione dei Monopoli di Stato, è stata acquistata dalla British American Tobacco. Questa azienda stranamente ha più di uno stabilimento sul territorio nazionale, tra i quali uno a Lecce. I dati forniti alle maestranze dai sindacati evidenziavano che lo stabilimento di Lecce era fortemente penalizzato; era la struttura con le peggiori *performance* economiche; viceversa, quello di Rovereto aveva la massima redditività. È sembrato quindi molto strano che un'azienda vada a chiudere l'unico ramo aziendale sostanzialmente in attivo. Gli stessi sindacati sembra abbiano ipotizzato fortissime ingerenze da parte di ambienti governativi dell'Unione. Parlando in questi termini, e ricordando che Lecce, tra l'altro, è anche il collegio elettorale del ministro D'Alema, viene da pensare che l'operazione non si è svolta nella massima trasparenza e regolarità.

che lascia tanti dubbi, e anzi quasi la certezza che una componente del Governo Prodi si sia frapposta alle scelte aziendali, al punto da far chiudere uno stabilimento in attivo per far rimanere aperto, viceversa, uno stabilimento fortemente in *deficit* e in crisi occupazionale.

e che, anche in virtù di questo, hanno acquisito nuove patologie di tipo sanitario. Sono donne impegnate su tutti i fronti, donne che lavorano e che rappresentano il centro vitale delle famiglie, giovani donne che crescono e vedono passare gli anni senza che siano tenute in alcuna considerazione quelle differenze di genere a livello sanitario che l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiaramente definito. Le donne, infatti, hanno caratteristiche fisiche ed esigenze di salute non ancora riconosciute come sarebbe loro dovuto e necessario. L'Organizzazione mondiale della sanità nel 1974 ha definito la salute come uno stato di benessere fisico, psichico e relazionale. Di conseguenza, nel momento in cui uno di questi tre elementi è alterato, si può rilevare lo stato di malattia. In questa ottica, la salute femminile deve essere sempre più oggetto di un'attenzione politica e sociale. L'evoluzione civile della società vede aumentare ogni giorno il numero delle donne che raggiungono la prima linea anche in campo lavorativo. un inevitabile aggravamento di situazioni di *stress*, che concorrono all'usura delle risorse psicofisiche, che le donne devono utilizzare anche sul fronte familiare. Il doppio lavoro, la propensione femminile ad occuparsi prima dei bisogni e della salute degli altri e poi dei propri, un interesse per la salute femminile prevalentemente circoscritto agli aspetti riproduttivi, la limitata partecipazione delle donne agli studi clinici sui nuovi farmaci: sono tutti fattori che dimostrano come le donne siano ancora svantaggiate rispetto agli uomini nella tutela della loro salute. Oggi, dunque, vogliamo ripartire da lei e ci poniamo subito una domanda: l'attuale sistema di assistenza sanitaria in Italia discrimina le donne? A dire il vero, questo non si può dire ma è vero che esistono diversi fattori determinanti uno stato di sostanziale svantaggio delle donne in tema di tutela della salute. Interrogarsi sul rilievo attribuito alla tutela della salute della donna significa rispondere anche ad un secondo quesito di base. La donna, come tale, necessita di un'assistenza sanitaria specifica e complessiva o è sufficiente ritagliare spazi settoriali mirati al sostegno delle esigenze sanitarie del mondo femminile? A ciascuna di queste due opzioni corrisponde non solo un modo diverso di concepire la salute della donna e dell'universo dell'assistenza sanitaria ma anche un diverso modo d'interpretare e valutare la programmazione e la normazione in ambito sanitario. Nella programmazione sanitaria nazionale emerge la mancanza di un approccio scientifico ai temi della salute femminile mentre nella politica legislativa più settoriale emerge in ambito emerge in ambito parlamentare una particolare attenzione al tema. Speriamo che da questo punto di vista noi possiamo invertire questa marcia. Sempre l'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme perchè le donne risultano sempre più svantaggiate rispetto agli uomini per tutto quanto riguarda la loro salute. Non c'è rispetto delle differenze di genere e non si tiene conto del fatto che appartenere ad un sesso rispetto ad un altro influenza la salute e la percezione stessa di questa. Non c'è consapevolezza, spesso da parte delle donne stesse, le quali sono le prime ad occuparsi della salute della famiglia trascurando la propria. In un documento molto bello del Dipartimento per la salute della donna, si evidenzia l'importanza e la complessità del tema della diversità femminile, sottolineandone l'ancora sostanziale misconoscenza e sottovalutazione. Sempre più, oggi, appare evidente che la ricerca medica è sempre stata condizionata dal genere. Gli argomenti scelti, i metodi utilizzati e la successiva analisi dei dati Il pregiudizio di genere è evidente non solo nella scelta dei temi, ma anche nel disegno di molte ricerche. Nei casi in cui le stesse malattie colpiscono uomini e donne, molti ricercatori hanno ignorato le possibili differenze tra i sessi per quanto riguarda gli indicatori diagnostici, i sintomi, la prognosi e l'efficacia relativa dei trattamenti differenti. Fin quando i ricercatori considereranno gli uomini come la norma, la cura medica offerta alle donne continuerà ad essere compromessa. In conclusione le donne sono più esposte ad alcune patologie, sono curate meno bene e molto spesso, con farmaci non sperimentati direttamente su di loro. Più di recente, il *report* annuale dello IOM (*Institute of Medicine*) ha rilevato nelle proprie conclusioni che la differenza di genere apre interrogativi su molte problematiche che finora non sono state neppure immaginate. La salute della donna è cambiata anche perché è cambiato il suo ruolo sociale. Oggi la donna è *overcommitted*, si confronta, cioè, con un carico di impegni maggiore rispetto a quelli che è in grado di gestire; molte donne devono fare i conti con la fretta, con una maggiore ansia, con un aumento dello stress e con i disturbi correlati. I disturbi psichiatrici sono in netta prevalenza femminili e le malattie cardiocircolatorie sono diventate la prima causa di morte delle donne. Il detto comune per cui l'infarto era definito come la malattia malattia che rende vedove, oggi non vale più. Adottare quindi in campo medico una prospettiva di genere e ridisegnare la ricerca come strumento di conoscenza che è alla base delle politiche sanitarie è una necessità e un passo fondamentale per pensare ad una salute anche a misura di donna. La prima volta in cui in medicina si parla della «questione femminile», e quindi di medicina di genere, risale al 1991, quando l'allora direttrice dell'Istituto nazionale di salute pubblica americano, Bernardine Healy, in un famoso editoriale della rivista «*New England Journal of Medicine*» parlò di «*Yentl Syndrome*» in riferimento al comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti del sesso femminile. Storicamente quando venivano messi a punto nuovi studi clinici, in particolare quelli relativi all'impiego di nuovi farmaci, venivano coinvolti soggetti di sesso maschile. Questo è stato per lungo tempo giustificato attraverso varie argomentazioni: difficoltà nell'arruolamento e nel mantenimento delle donne negli studi clinici; preoccupazioni riguardo alle interferenze indotte dalle variazioni ormonali tipiche dell'organismo femminile sull'effetto delle sostanze farmacologiche da testare; preoccupazioni circa la possibilità di esporre a rischi di tossicità donne potenzialmente fertili. Sfortunatamente se un farmaco o un presidio medico-chirurgico non è espressamente testato sulle donne, non esiste modo di conoscere quali saranno le reali condizioni di efficacia e di sicurezza su di loro. Infatti in medicina, efficacia e sicurezza si misurano attraverso parametri che sono fortemente correlati a fattori come l'età, il sesso, le caratteristiche e la composizione dei tessuti e, a loro volta, sono associati in maniera specifica alle caratteristiche biologiche legate al sesso, come agli ormoni o alla prevalenza nei due sessi di particolari caratteristiche (corporatura, stili di vita, concomitanza di disturbi e così via). In definitiva, allora, cosa si sta facendo per la costruzione di una «medicina di genere», cioè di una medicina che tenga conto delle fisiologiche differenze tra uomini e donne sia nella teoria che nella pratica clinica? All'avanguardia ci sono gli Stati Uniti: alla Columbia University di New York è stato recentemente organizzato un corso specifico di medicina di genere; in Svizzera è nato da tempo un corso di laurea specifico presso la facoltà di medicina. La Comunità europea, seppur con molti anni di ritardo, fin dal 1998 ha incluso all'interno dei programmi di ricerca un invito alle donne a partecipare e a presentare progetti. Oggi si sta cominciando a rendere fattiva anche questa ipotesi.

al meglio che c'è su questo in Europa e nel mondo. Chiediamo che almeno già da quest'anno si possa partire con un corso di specializzazione, un *master* *post* laurea o *post* specializzazione, e che da subito poi possa iniziare anche l'*iter* della costruzione di un percorso specialistico, così come accade in Svizzera. Lo chiediamo perché in Italia ci sono professionalità, perché ci sono già ospedali, ci sono professionisti che, da questo punto di vista, stanno creando un'ottica nuova e crediamo che questo Parlamento e questo Governo possano veramente dare, con una chiave di volta, un'inversione, una prospettiva straordinaria e accogliere questa grandissima sfida. Concludo ringraziando la senatrice Serafini

ringrazio anch'io la senatrice Bianconi e tutti coloro che hanno sottoscritto la mozione di cui è prima firmataria, così come le colleghe e i colleghi di Rifondazione Comunista e la senatrice Valpiana. È un ringraziamento non formale perché le argomentazioni che sono presenti nelle mozioni hanno dei punti di contatto molto forti. Scegliere oggi di introdurre in medicina il principio della differenza femminile rappresenta ben più che una questione esclusivamente biologica o di uguaglianza tra generi, rappresenta una questione squisitamente politica che definisce un'altra tappa del cammino delle donne che parte dall'esperienza concreta, prima fra tutte quella della propria corporeità. Alain Touraine, in un libro appena uscito in Francia: «*Le monde des femmes*» traccia le linee di tale ragionamento. Il testo è estremamente significativo perché è frutto di un percorso di ricerca attraverso gruppi di discussione con donne di diversa origine ed estrazione sociale. Touraine afferma che alla domanda: «chi siete?» le donne rispondono oggi: «sono una donna, mi costruisco come donna e lo faccio a partire della mia corporeità». Touraine critica la visione meccanica del concetto di genere e lo fa mettendo in rilievo l'esperienza vissuta a partire da quella corporea. Dice Touraine: «L'idea di genere porta con se una sorta di determinismo sociale e anche ideologico della condotta femminile, così la loro soggettività non è altro che un insieme di riflessi e di illusioni che rischiano di non renderle più capaci di un'azione autonoma. Al momento in cui si sostituisce a questo vago determinismo la tesi più precisa del dominio maschile, bisogna prendere coscienza di tutto ciò che non è stato considerato: la storia personale, l'emotività, le relazioni interpersonali, in sintesi tutto ciò che occorre alla formazione della personalità». Perciò non bisogna scegliere fra determinismo sociale e una soggettività di solo ordine psicologico. Il corpo, quindi, è il veicolo dell'esperienza reale e quindi i metodi e i criteri d'intervento su di esso divengono fondamentali per la costruzione del sé cui le donne oggi tendono, proprio secondo l'indagine condotta da Touraine. La divisione tradizionale dei ruoli tra i generi è stata sottoposta, negli ultimi decenni, a profondi mutamenti. Non c'è settore della società, dall'economia alla politica, dalla cultura alla famiglia, che non sia stato investito dall'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Tuttavia, la struttura della società, le sue gerarchie, le sue priorità, i suoi punti di vista hanno difficoltà a recepire pienamente questo cambiamento. Ne conseguono, spesso, sottovalutazioni e ritardi nel comprendere le contraddizioni che ne scaturiscono. Le modalità di rappresentazione e identificazione dei ruoli sono ancora influenzate dai modelli culturali tradizionali e questi influiscono non poco sul modo in cui le donne e gli uomini sono in grado di percepire se stessi ed il proprio ruolo e di vivere con piena consapevolezza le implicazioni insite in questa fase di trasformazione. Lo stesso terreno della salute e del benessere è attraversato da problemi ed inquietudini inediti, non sempre colti in modo adeguato. La messa in evidenza dei tratti della salute delle donne costituisce un contributo rilevante a comprendere tale trasformazione, nonché a sperimentare misure efficaci per rispondere ad alcuni bisogni specifici di cura sia delle donne sia degli uomini e a porre in relazione salute delle donne e salute dei bambini. Tra i mutamenti generali va segnalato il passaggio da una famiglia di tipo plurinucleare ed estesa ad una di tipo mononucleare e ristretta. I dati ci dicono che l'Italia è il Paese con il più basso quoziente di natalità d'Europa,

Il recente positivo innalzamento del tasso demografico in Italia è quasi esclusivamente riconducibile all'iscrizione all'anagrafe di bambini immigrati. Le donne italiane non rifiutano la maternità, tutt'altro. C'è un divario molto elevato tra maternità desiderata ed effettivamente realizzata.

Questo comporta, oltre all'esplicito rinvio dell'esperienza della maternità, una forte compressione del periodo fecondo in un arco temporale di pochi anni, nel quale mettere al mondo più di un figlio è diventata l'eccezione piuttosto che la regola. L'Italia condivide, con pochissimi altri Paesi europei, il più basso tasso di occupazione femminile. Nella ricerca ISTAT del 2003, il tasso di occupazione femminile in Italia risulta essere del 42,7

L'Italia è un Paese caratterizzato da uno scarso interesse per le politiche di conciliazione tra i tempi della vita e i tempi del lavoro. Il tema della conciliazione deve essere visto soprattutto in riferimento alla qualità della vita. Sempre secondo i dati ISTAT del 2002, il 50,4 per cento delle donne con bambini piccoli lavora 60 ore o più alla settimana, tra lavoro esterno remunerato e lavoro in famiglia non remunerato. E' indicativo che in Italia il 20 per cento delle madri con un lavoro all'inizio della gravidanza, ad esempio, dopo circa 18-21 mesi non ha più lavoro, mentre il 36 per cento di quelle che hanno continuato a lavorare dichiara di avere problemi molto seri nel conciliare l'attività lavorativa e gli impegni familiari. L'assenza di incisive politiche di conciliazione e gli impegni sempre maggiori richiesti alle donne hanno di conseguenza portato ad un aumento dello *stress*; le donne sono più colpite da depressione, attacchi di panico, ansia sociale, disturbi del comportamento alimentare. Patologie, che in passato colpivano maggiormente la popolazione maschile, quali le malattie cardiovascolari ed alcuni tumori, come quello al polmone, stanno diventando importanti cause di morte nell'universo femminile. Anche la presenza di un'importante componente femminile nei flussi migratori, circa il 49,9 per cento della popolazione immigrata, pone delle istanze nuove ai servizi socio-sanitari anche in relazione a pratiche di mutilazioni genitali femminili e alle diverse tradizioni culturali. Criterio fondamentale deve essere quello del pieno rispetto dell'autonomia e della dignità delle donne. Il rapporto dell'UNICEF del 2007 è dedicato ai diritti delle donne e al legame esistente tra essi e gli effetti positivi per la loro salute e la nutrizione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione dei loro figli. Il corpo e la salute della donna sono un tema fondamentale della costruzione dell'uguaglianza di genere. Questi due elementi sono, da sempre, terreno di negazione o affermazione di tale uguaglianza. Come ha sottolineato la Conferenza mondiale ONU sulle donne del 1995 «La violenza alle donne è la manifestazione della storica differenza in termini di potere all'interno delle relazioni di genere». In Italia, oltre 14 milioni di donne sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita, senza esclusione dello stato di gravidanza ed il 69,7 per cento degli stupri sono perpetrati dal proprio *partner*. Ciò determina effettivi traumi fisici e psicologici rilevanti che incidono profondamente anche sulla dinamica del rapporto tra donna e bambini e bambine, asse fondamentale per l'Agenda del millennio richiamato dal rapporto UNICEF 2007. Molti studi dicono che la violenza sulle donne non è mai reazione ad un torto e non è neanche soltanto lo sfogo maschile a proprie insoddisfazioni, frustrazioni. È molto di più e richiama un livello qualitativamente diverso; attiene a profonde motivazioni culturali, ai modelli del rapporto tra i generi, tra le persone. La violenza, sia quella morale, psicologica, fisica, economica e sessuale, da parte del *partner* è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo cui sono connessi privilegi e soprattutto di un ruolo gerarchicamente dominante. La violenza diventa quindi uno strumento usato contro la donna che non vuole riconoscere questo potere, questa gerarchia nei rapporti, così come ci è stata consegnata dal passato. Forse per questo la violenza non si ferma neanche di fronte alla gravidanza. Le donne che subiscono violenza e spesso i loro figli, in virtù degli attacchi subiti, appaiono deboli, svuotati, «senza sogni», come è scritto in un bel documento del Centro antiviolenza di Udine. Chi non ha maturato culturalmente e dal punto di vista del metodo le cause dei centri antiviolenza sulle donne potrebbe essere indotto a puro pietismo. All'opposto, la debolezza va considerata uno stato momentaneo provocato da un attacco subìto. Questa competenza è stata maturata attraverso l'accoglienza concreta di tantissime donne, il lavoro e le competenze di prim'ordine di psicologhe, assistenti sociali, psicoanaliste, avvocate, insegnanti e magistrate. Investire sulla salute delle donne comporta non solo un'azione diretta sulla loro salute, ma può determinare un significativo miglioramento della condizione di salute dei bambini e degli adolescenti e, conseguentemente, delle condizioni di salute delle future generazioni. Il benessere delle donne ha pertanto una diretta influenza sul benessere dei bambini. L'adolescenza per le ragazze è un periodo di particolari cambiamenti, sia dal punto di vista fisico sia psichico, che necessita di forme di attenzione e di informazione adeguate. Invece cosa succede? C'è una protezione o siamo in presenza di una vera e propria mancanza di protezione fino alla distorsione dei bisogni delle adolescenti e delle giovani donne? Il CENSIS, nell'indagine di quest'anno, propende per la seconda ipotesi, sottolineando che «d'altra parte sono corpi di donne giovani quelli esibiti in modo compulsivo sui *media* e sono evidentemente proprio le ragazze, nella fase in cui si conclude il loro percorso di maturazione, ad essere più vulnerabili sotto questo profilo. Anche questo andamento viene confermato dai dati e sono infatti con maggiore frequenza le più giovani a vedere nelle donne che appaiono in televisione anche modelli realistici, nei quali è possibile identificarsi e da ritenere che, anche se artificiali, i modelli mediatici sono quelli a cui la maggior parte delle donne vorrebbe somigliare». Il CENSIS ritiene che le conseguenze siano rilevanti per la salute psicofisica delle donne «in questo scenario risulta dunque di particolare interesse verificare come e in quale misura l'analisi delle percezioni, delle opinioni e dei comportamenti delle donne italiane, nella sfera del rapporto con se stesse e con le immagini, registri questa pressione mediatica sui loro corpi, e se ne emergano rischi in termini sociali Dello stesso avviso è Umberto Galimberti che, in un bel saggio, mette in relazione questo modo di considerare il corpo femminile ad una espropriazione delle donne medesime. Egli si chiede: «Ma dove parla il mondo femminile, dove si descrive, dove si racconta? Certamente non nei giornali femminili che riempiono le nostre edicole. Lì a parlare è la moda, come se le donne facessero dipendere la loro identità dai vestiti, la bellezza che tutte, se non per natura, almeno per artificio, dovrebbero raggiungere, la dieta perché esiste anche un'accettazione sociale che privilegia lo stile anoressico, la cucina perché gli uomini si prendono anche per la gola, la salute in modo che palestre, farmacie ed erboristerie possano speculare vendendo mezze bugie e mezze verità, e infine la sessualità dove l'immaginario mette in scena il suo teatro di angosce e di desiderio chiamando a raccolta in modo sfuso e confuso tutti i sogni diurni e notturni. Tutto ciò non è il mondo femminile, ma sfruttamento di quel mondo, che ancora una volta si chiude, cupo su se medesimo, anche se in superficie danzano tutti i colori della carta patinata per celebrare quel santuario ideologico che è diventato ai nostri giorni il corpo, reso inespressivo da cerimoniali proprio che lo esaltano». In molti Paesi con sistemi sanitari sviluppati, compresa l'Italia, si è assistito ad un progressivo aumento della frequenza di procedure diagnostiche e terapeutiche complesse ed invasive estese a gran parte delle gravidanze. Non si è sviluppata un'adeguata iniziativa per favorire la preparazione al parto e per l'assistenza dopo il parto, con particolare attenzione alle forme di depressione *post partum*. Esistono forme di disagio, che colpiscono in particolare donne immigrate, che possono portare all'abbandono dei bambini appena nati. La salvaguardia dell'interesse superiore del minore e del rispetto della dignità delle donne sollecita un punto di vista non persecutorio. Questa medicalizzazione dell'evento nascita, spesso non necessaria dal punto di vista clinico, oltre ad indurre un aumento dei costi, ha determinato un incremento dei rischi di problemi iatrogeni ed in generale una ridotta qualità delle prestazioni sanitarie. È opportuno che la medicina assuma complessivamente il principio tecnico-scientifico

La crisi deriva da una impostazione che non sa porre correttamente a confronto i problemi di salute delle donne con quelli degli uomini. In tal senso la conservazione del sangue del cordone ombelicale può costituire, anche per la ricerca, un ponte che parte dalle donne e arriva agli uomini e ai bambini; l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha costituito dal 2002 il Dipartimento per il genere e la salute della donna con la costituzione di questo dipartimento l'OMS riconosce che esistono differenze nei fattori che determinano la salute e nei fattori che determinano il carico di malattia per uomini e donne;

Il Dipartimento della salute americano ha costituito nel 1991 l'Ufficio sulla salute della donna, così come un documento dell'Organizzazione mondiale della sanità evidenzia come il pregiudizio di genere sia evidente non solo nella scelta dei temi, ma anche nel disegno di molte ricerche. La prima volta in cui in medicina si parla della questione femminile e quindi di medicina di genere risale al 1991, in riferimento al comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti del sesso femminile. In Italia, nell'ambito degli studi universitari, in particolare nella facoltà di medicina e chirurgia, non si è fatto ancora nulla per la costruzione di una medicina di genere, cioè di una medicina che tenga conto delle fisiologiche differenze tra uomini e donne sia nella teoria che nella pratica clinica. Gli Stati Uniti sono all'avanguardia, come si vede alla Columbia University di New York. In Svizzera è nato da tempo un corso di laurea specifico presso la facoltà di medicina. La Comunità Europea, seppur con anni di ritardo, ha incluso all'interno dei programmi di ricerca un *focus* sulle donne. Nel 1999 l'Italia ha visto la nascita del gruppo di lavoro «Medicina Donna Salute» che ha dato un contributo fondamentale all'individuazione di una specifica problematica di genere. Nel 2005 è nato l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che si occupa della salute della donna con una visione a 360 gradi. Infine, nel novembre del 2005 è nato il progetto «La salute delle donne» presso il Ministero della salute nell'ottobre del 2006, sempre nell'ambito del progetto «La salute delle donne», è stato avviato lo «Studio della medicina di genere attraverso il sistema di monitoraggio delle dimissioni ospedaliere». Al fine di rafforzare tali iniziative e sviluppare un'azione conseguente, è necessario (come ha detto la collega Bianconi e come si evince nella mozione presentata dalla collega Valpiana) istituire, alla stregua di quanto è stato fatto in America e in Svizzera, un corso di specializzazione in medicina di genere.

tenere presente il punto di vista di genere come una delle linee guida del Servizio sanitario nazionale e coinvolgere la rete dei Centri antiviolenza delle donne in un'opera di monitoraggio e prevenzione della violenza alle donne, in modo particolare durante ed immediatamente dopo la gravidanza. occorre favorire forme reali di accoglienza, rifuggendo ogni spirito persecutorio, per le donne in difficoltà che sono costrette ad abbandonare il proprio bambino in luogo sicuro per l'integrità della salute e del benessere del bambino stesso. Colleghe e colleghi, mi avvio alla conclusione. In questi anni molti aspetti della vita delle donne sono cambiati ma i rapporti tra i sessi faticano ad essere rapporti tra eguali. Spesso il confine tra le diverse forme di violenza è molto sottile: talvolta la stessa «dipendenza amorosa», se non è tra eguali, può esprimere autosvalutazione, che può aprire la strada ad una qualche forma di violenza.e a forme gravi di depressione. Norwood, nel libro «Un pensiero al giorno per donne che amano troppo», afferma: «Non si è mai troppo intelligenti, troppo belle, troppo affascinanti, troppo ben educate, troppo ricche, troppo istruite, troppo dotate o troppo di successo per amare troppo. Nessuna di queste condizioni ci libera del tutto o in parte dal rischio di contrarre dipendenza relazionale o, se è per questo, da qualsiasi forma di dipendenza». Chi decide di interrompere la dipendenza, come afferma in un suo precedente libro, invece di una donna che ama qualcun altro tanto da soffrirne, sarà una donna che ama abbastanza se stessa da non voler più soffrire. L'unica sofferenza da augurarci, quindi, colleghi e colleghe, e da augurare anche agli uomini sarebbe quella descritta da Platone nel «Simposio»: "L'amore non fa né subisce ingiustizia, sia fra gli dei che fra gli uomini. Poiché lui non soffre per forza quando gli accade di soffrire; perché la forza non tocca l'amore. E quando agisce non agisce con forza; perché a ciascuno acconsente a obbedire in tutto all'amore".

Possiamo salutarla e rivendicarla come una conquista dell'onda lunga del femminismo, una conquista che viene da lontano perché i tempi della storia sono lunghi e la pazienza attiva è una virtù. II rapporto tra donne e medicina, donne e scienza non è un rapporto facile, non lo è per quelle che esercitano scienza e medicina e non lo è per le donne utenti, per quante usano saperi e servizi e vorrebbero essere soggetti e non oggetti parcellizzati agiti da altri. Non lo è ora e ancor meno lo è stato in passato. Pertanto, a proposito di donne, salute e medicina, è difficile non andare con la memoria alle antenate, le erbarie, guaritrici e levatrici, e se è vero che la storia non si fa con i se, nulla ci impedisce però di provare per come sono andate le cose e per gli esiti che avrebbero potuto avere se fossero andate diversamente, se non vi fosse stata quella rottura drammatica che va sotto il nome di caccia alle streghe. Si giocò allora una partita simbolica sulla sessualità, quella femminile, proprio nella definizione dei tratti, i comportamenti e i patti attribuiti alle donne che vennero considerate e condannate come streghe. Le donne accusate di stregoneria erano portataci di un sapere popolare, radicato e diffuso, fondato sull'esperienza, un sapere che fino al Medioevo era accettato come parte del sistema simbolico e culturale del tempo e che, invece, con il Rinascimento e con la riorganizzazione del pensiero scientifico, venne escluso dall'ufficialità. Il famoso *Malleus* *maleficarum* (il martello delle streghe) del 1486 è, da questo punto di vista, uno scritto fondamentale perché rappresenta (la descrizione di cosa sia e cosa faccia la strega) il compimento di un processo cruento di rottura, di espropriazione e di scontro iniziato con l'Inquisizione. Nei secoli dell'Alto Medioevo l'*herbaria*, cioè l'esperta di erbe, era la curatrice, quella che esercitava una medicina povera, legata al saper fare. In tutto il Medioevo l'ambito nel quale le donne dominavano incontrastate è quello dell'ostetricia e della ginecologia. Nel XIII secolo i trattati di medicina parlano del taglio cesareo, pratica che era appannaggio esclusivo delle ostetriche, ma, nello stesso tempo, si istituzionalizza e si regolamenta la professione medica e si diffonde il divieto di accesso nelle nuove facoltà di medicina alle donne. La cacciata dalla professione si trasforma successivamente in una caccia vera e propria: le donne medico vengono processate con l'accusa di esercitare pratiche magiche; per secoli ciò che non aveva suscitato diffidenza, paura, diviene pericoloso. Sempre nel *Malleus maleficarum*, un secolo dopo, il percorso si è ormai compiuto e così si affermerà che «nessuno nuoce alla fede cattolica più delle ostetriche» e che dovrà ritenersi strega «la persona che libera da malefici e guarisce da malattie senza conoscere la medicina», cioè la donna che opera fuori dal controllo delle istituzioni esercitando un potere frutto di un sapere che può produrre libero pensiero e conoscenza. Queste donne vengono bruciate insieme agli eretici. Le vittime furono tante, centinaia di migliaia, un vero e proprio femminicidio, come si dice adesso. Erano prevalentemente levatrici, accusate di aiutare a partorire, di aiutare ad abortire, di conoscere mezzi anticoncezionali, di essere guaritrici e di essere ovviamente di facili costumi. Con questo scontro, ovviamente uno scontro di classe e di sesso durato quattro secoli, si tolse di mezzo, insieme alle donne, anche una medicina popolare ed in particolare un sapere ostetrico-ginecologico che era tutto nelle loro mani. Penso che il cerino sia sempre acceso e mi domando se oggi qualcuno questo cerino in mano lo stia tenendo. La storia comunque è lunga. La professione medica si strutturò poi in modo sempre più gerarchico: il dottore in cima alla piramide e farmaciste, cerusiche e chirurghe, istruite da mariti e genitori, organizzate in corporazioni, preparavano ricette, salassavano o operavano. Si deve arrivare alla seconda metà dell'800 perché in Italia alle donne si riaprano le porte di licei ed università. Se facciamo un salto di almeno un secolo, è al femminismo del nostro tempo che si deve la forte ripresa dei temi legati al corpo, alla salute, all'autodeterminazione: la coscienza che non si dà libertà femminile senza signoria sul proprio essere corporeo. Negli anni '60, negli Stati Uniti, le femministe, insieme alla pratica politica dell'autocoscienza, il partire da sé in quanto donne, con specifici bisogni e desideri, misero in discussione ruoli sociali e ruoli sessuali imposti, in primo luogo la famiglia, la sessualità subordinata al piacere maschile; diedero vita a gruppi di *self-help* nei quali si provava a condividere, anche attraverso le auto-visite, competenze, vissuti, informazioni relative al corpo ed alla sessualità, con l'idea di riappropriarsi di un sapere personale perduto a causa della medicalizzazione del corpo e di eventi naturali come il ciclo mestruale o il parto.

In Italia, nei mitici anni '70, i temi della salute, del corpo, della sessualità, del rapporto delle donne con la medicina e le istituzioni diventarono elaborazione centrale di parte del movimento femminista. Donne del movimento, in particolare a Torino, diedero vita ai centri di salute e di medicina delle donne. Il punto di partenza fu la considerazione che molte funzioni fisiologiche femminili, in particolare quelle legate alla sfera della riproduzione, erano trattate come stati di malattia e per questo delegate al medico. La messa in discussione dei princìpi che regolavano le nascite, quali il divieto alla contraccezione e il divieto di aborto, erano immediatamente in conflitto con la politica e con la morale allora imperante, cioè ogni espressione di bisogni e desideri di bisogni e desideri delle donne rappresentava una minaccia al sistema di controllo sul corpo delle donne. Quella di quegli anni è stata la stagione da cui sono scaturiti grandi cambiamenti, una vera rivoluzione per certi versi: ricordiamo il nuovo diritto di famiglia, il divorzio, l'istituzione dei consultori, la contraccezione e l'aborto. In questi 30 anni la riflessione non è cessata, si è estesa al rapporto tra donne e scienze, alle conseguenze materiali, culturali e simboliche dell'impiego delle biotecnologie, come ci ha mostrato l'esito del *referendum* sulla legge n. 40. Molta strada comunque è stata fatta, molta deve esserlo ancora e la discussione di oggi ci indica una direzione di lavoro precisa con l'obiettivo prioritario di diminuire le disuguaglianze nei confronti della salute, nello specifico quelle di genere. Mettere al centro la medicina di genere non è solo la sensibilità alle specifiche condizioni di salute o al ciclo biologico delle donne: è riflessione sulla parzialità della scienza e sulla sua pretesa di neutralità; è mettere al centro la persona sessuata; è interrogarsi sulla relazione medico-paziente e su come sono concepiti i corpi dalla scienza, come aggregati di organi e funzioni poiché non rientrano nell'osservazione medica e nei protocolli di ricerca corpi che abbiano sentimenti, percezioni, parole, capacità di autoconoscenza.

malattia. Questo significa affermare una concezione complessiva della salute, capace di coniugare i fattori individuali, biologici e psicologici con fattori psico-sociali ed ambientali, quindi, per esempio, limitare la convinzione che la salute delle donne sia prevalentemente influenzata dalle vicende del ciclo biologico. La conseguenza di questa convinzione è un pregiudizio individuabile in una serie di mancanze nella prospettiva della ricerca e della clinica: per esempio, la mancanza di indagini sui fattori di rischio nelle varie patologie, collegati alla vita delle donne, in particolare al sovraccarico lavorativo e le varie forme di violenza; per esempio, la mancanza di definizione di pratiche diagnostiche e terapeutiche non valutate solo sul modello indifferenziato maschile; per esempio, la difficoltà di costruire profili di rischio femminile per la mancata raccolta dei dati disaggregati per sesso; per esempio, la mancata valutazione della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza femminile. Come detto, l'Organizzazione mondiale della sanità nel 2002 ha costituito il Dipartimento per il genere e la salute della donna. Con questo atto si riconosce che esistono differenze nei fattori che determinano la salute e la malattia per uomini e donne. Le differenze di genere tra uomini e donne si riferiscono - i cosiddetti determinanti socio-economici - a dati culturali e sociali. Le donne vivono in condizione di minori risorse, minore occupazione, minori livelli occupazionali, maggiore carico di lavoro e maggiore violenza rispetto agli uomini. E ciò si riflette sulle loro condizioni di salute. per modificare e migliorare la qualità della salute bisogna agire, oltre che sui servizi della salute, anche sul contesto socio-economico e sugli stili di vita che a questo sono legati. Nel piano presentato a marzo dalla signora ministro Turco per la promozione e la tutela della salute delle donne sono previste molte azioni puntuali. Credo che sia importante sottolinearne una, che è anche centrale

così come nel programma dell'Unione, così come richiesto nelle nostre mozioni, sarà una scelta prioritaria, potremmo evitare di ridurre tanta incapacità nell'affrontare sé stessi ed il futuro. I consultori sono un aspetto importante della lotta delle donne, come dicevo prima.

dall'ascolto delle operatrici, dalla presenza delle donne e dalla discussione delle varie situazioni ed è sempre stato visto come un patrimonio unico da non disperdere, nonostante tutti gli elementi critici che ci sono stati dalla fine degli anni '80 proprio per quelle situazioni di carenza e di attribuzione della missione del consultorio. L'accento sull'importanza di allestire servizi per la salute primaria - servizi caratterizzati da un approccio integrato, secondo un modello sociale di salute sostituito da una modalità operativa basata sull'offerta attiva, operanti mediante la relazione di comunicazione orizzontale -

dall'Osservatorio per la salute delle donne, costituito nel 2003 dall'amministrazione comunale di Torino, dal Coordinamento per l'autodeterminanzione delle donne della Casa delle donne di Torino e dal Centro studi storici delle donne dell'Università di Torino. Questi tre soggetti insieme

poi recuperata all'interno del piano sanitario della Regione Piemonte, proprio perché si era costituito questo rapporto virtuoso tra vari soggetti e perché tale realtà,

nel corso della loro storia e del loro lavoro, hanno affrontato più direttamente e in maniera più partecipata tali problematiche. Nella nostra mozione è presente un aspetto che è stato sollevato anche nelle altre mozioni, quello dell'istituzione, così così come in altri Paesi, di un corso di specializzazione post‑laurea in medicina di genere. Ci sembra molto importante fare questo salto di qualità, valorizzando molto i contenuti che già in qualche modo si sono prodotti e dandogli una una veste definita ed istituzionalizzata. C'è ancora un argomento che non abbiamo affrontato, che però mi sembra utile, cioè la condizione di quante donne a vario titolo lavorano nelle istituzioni sanitarie e negli ospedali piuttosto che nelle residenze per gli anziani. Il potere medico maschile è ancora molto forte. È interessante conoscere e capire quali sono le condizioni di lavoro e le condizioni di carriera, non soltanto nel senso verticale

È sempre forte la discriminazione nei confronti delle donne, perché, oltre alla vita lavorativa, hanno anche una vita affettiva intensa e un carico che rivendicano di poter rivendicano di poter gestire. Credo allora che un'altra linea di indagine quando si parla di medicina delle donne debba tener presente le operatrici del settore, per capire cosa accade e quali sono i meccanismi che si possono mettere in atto per produrre effetti positivi. Termino qui il mio intervento; aspetto le risposte e spero, come è già stato detto, che con queste mozioni si dia luogo ad un impegno concreto, duraturo e fattivo, che ci veda in altri momenti a discutere i dati, a monitorare

Non è un caso: il punto di vista femminile, in particolar modo sulla salute, ma non solo, non è frutto di un femminismo ideologico o di una cultura autoreferente limitata ad alcune *élite* femminili, ma invece di una rivoluzione profonda, la più pervasiva, positiva e tuttora vitale che ereditiamo dal secolo passato, quella delle donne. Si tratta di una presa di coscienza fortemente ancorata all'esperienza differente dell'essere donna nella sfera simbolica e in quella sociale. La differenza, iscritta nel corpo femminile, è all'origine della fondazione di una nuova soggettività morale che ha attraversato ogni campo del sapere modificando statuti e assetti disciplinari. La proposta, congiuntamente avanzata al Governo, di istituire, come già si è fatto in altri Paesi, un corso di specializzazione in medicina di genere, così come quella di dare vita a un osservatorio sul benessere e la salute delle donne, non è da intendersi come pura aggiunta affiancamento alle altre specialità o ad altri osservatori. Quando parliamo di donne parliamo di uno dei due sessi che è all'origine della specie ed è, tra i due, quello maggiormente impegnato nella riproduzione della specie stessa e, dunque, della necessità che la medicina sappia contrastare ogni pretesa di scientificità neutra valida in tutti i casi, indifferentemente, per uomini e donne, al fine di raggiungere mete e traguardi sempre più significativi nella cura e nella prevenzione di malattie che differentemente colpiscono l'umanità maschile da quella femminile. Sembrerebbe persino ovvio nel campo della salute che la ricerca, la scienza clinica, i percorsi scientifici si debbano sviluppare coerentemente con i corpi e la vita reale e differente di donne e uomini; eppure, l'ovvio è il contrario. C'è la prosecuzione di attività indifferenziate, sia nei presupposti statistici, sia nei programmi e nelle azioni formative, che solo quando sono le donne a decidere assumono un punto di vista differente, cioè differentemente orientato alle donne e agli uomini reali. La nostra discussione parlamentare intorno a questi temi è dunque particolarmente importante e può avere ricadute significative sul piano sociale, implicando e intrecciandosi all'azione di Governo, a quella legislativa e incontrando certamente l'interesse di una vasta opinione pubblica. La storia della medicina a proposito delle donne è costellata di crimini; crimini non metaforici. Il parto cesareo vede la luce, per così dire, con un taglio contro la madre, la madre contro il bambino, *mors tua, vita mea*, in favore della vita del nascituro; ne parla molto bene la nostra collega, la senatrice Maria Luisa Boccia, in un bellissimo libro. È storia È storia sociale quella delle epidemie di setticemia puerperale, provocate dai ginecologi che, visitando in serie le puerpere, senza nemmeno lavarsi le mani, fino alla metà del secolo scorso, facevano così morire le donne. Senza volermi dilungare, mi preme invece esaltare l'opera del professor Veronesi, una straordinaria presenza italiana nel campo clinico e della ricerca medica, un vero amico delle donne, che si è opposto e si oppone all'idea ordinaria della mutilazione femminile per trattare la senologia oncologica sia dal punto di vista chirurgico che terapeutico e clinico. Tuttavia si tratta di un'eccezione; la normalità, ripeto, è un'altra. La classe medica, il mondo della ricerca, ma soprattutto i decisori, continuano ad essere più uomini che donne e questa è la differenza più corposa e visibile e non, invece, quella del corpo delle donne, con i suoi tempi, i bisogni, i sintomi, le patologie differenti che dovrebbero interrogare continuamente la medicina, la ricerca e la politica. Le donne vivono sei-otto anni in media più degli uomini e la differenza di genere si accentua anche con il progredire dell'età. Le donne più degli uomini fanno l'esperienza del deterioramento della propria capacità funzionale, a cominciare dai movimenti, e vivono il paradosso di essere più degli uomini soggette ad ammalarsi, ma contemporaneamente avere una mortalità più bassa. È incredibile come queste differenze siano costantemente osservate, soprattutto fortemente percepite socialmente e, tuttavia, ancora troppo poco studiate, al punto che non si sa ancora dire in che misura queste differenze siano da attribuire a fattori sociali piuttosto che biologici.

Oppure, gli uomini si ammalano di più per eventi cardiovascolari; tuttavia, quando le donne si ammalano, muoiono più facilmente. Perché? Dipende dalle procedure di diagnosi che sono meno sensibili per le donne? O piuttosto sono le terapie che sono meno efficaci? La professoressa Paola Muti, direttore scientifico dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena, intervenendo recentemente ad un convegno, svoltosi a Napoli e voluto dal ministro Turco, sulla salute delle donne, ha citato un recente studio spagnolo che ha studiato un vasto campione di 7.000 donne e uomini, ricoverati per infarto del miocardio acuto. Da questo studio risultava che nonostante donne e uomini fossero stati nella stessa misura sottoposti ad angiografia, poi, un numero molto inferiore di donne era stato riperfuso. Non solo, un numero ancora più basso di donne aveva ricevuto i trattamenti anticoagulanti, nonostante le linee guida a questo proposito fossero perentorie. Infine, anche nelle dimissioni delle donne, erano destinati un numero di presidi ridotto rispetto agli uomini. Tutti questi fatti si sono poi comprensibilmente tradotti in una più alta mortalità entro il ventottesimo giorno dall'infarto. La salute delle donne in concreto passa anche molto attraverso la collocazione centrale, il ruolo di sostegno e di cura della famiglia e delle relazioni familiari. Un recente studio dell'università di Padova ha mostrato come, in seguito ad una grave malattia che riguardi un figlio, è il 70 per cento delle donne che deve abbandonare il lavoro esterno per sopperire alle necessità di cura del figlio stesso. Questi dati così forti indicano come attraverso una nuova strutturazione dei *network* di cure primarie e di continuità assistenziali, indicate tante volte dal ministro Livia Turco, passi anche una nuova dimensione meno discriminante e di minore impatto sulla salute delle donne. In qualità di senatrice della Campania, una Regione del Sud che patisce una triste quantità di primati negativi a proposito della salute delle donne, sono particolarmente grata al ministro Livia Turco, che ha scelto, in occasione dell'8 marzo, di presentare a Napoli le linee di un piano di azione che assume proprio il diritto alla salute delle donne quale diritto forte, tale da promuovere e tutelare tutti gli altri diritti, sia sociali, sia civili e politici. Si tratta di un quadro di obiettivi strategici di azioni, in parte già significative e deliberate ed in parte da implementare, che effettivamente puntano a rendere la salute delle donne

al convegno di Napoli è stato dato ad alcune proposte, come per esempio uno spazio adolescenti all'interno consultori familiari, sportelli dedicati contro la violenza sulle donne su tutto il territorio nazionale, a cominciare dal pronto soccorsi, le modifiche della legge n. 53 sui congedi parentali per garantire più tempo a casa per genitori e bambini prematuri, così come il tema dell'educazione alla genitorialità e a campagne di prevenzione mirate sui tumori femminili hanno, nella nostra realtà campana, lasciato un segno profondo e positivo, rinnovando la speranza di cambiamento e la motivazione di tante donne: cittadine, operatrici della sanità, amministratici, donne delle istituzioni e della politica. Da molti anni tante donne delle associazioni e delle istituzioni sono impegnate e concentrate su una battaglia singolare; ci battiamo contro l'epidemia dei parti cesarei in Campania. Sì, epidemia. Nel 2003, a titolo di esempio, sono nati con taglio cesareo in Campania 34.330 bambini,

che parla del 20 per cento. Sappiamo che se fosse rispettato il ricorso fisiologico al cesareo, cioè avvicinandosi al 20 per cento, nello stesso anno avremmo avuto circa 23.000

si tratta solo del 12 per cento dei neonati. Certamente non è spiegabile con le caratteristiche delle madri il fatto che le donne assistite in strutture private, dove si concentra un basso tasso di rischio ostetrico, rischino per il 40 per cento in più delle altre donne con il ricorso al taglio cesareo. Molte e concrete proposte sono state avanzate in questi anni per il contenimento dei tagli cesarei. Oggi a quelle piattaforme che restano valide e riguardano i consultori, i centri nascita, il potenziamento degli organici delle ostetriche, abbiamo abbiamo trovato, come donne, la forza di aggiungere la costituzione di comitati ispettivi con la partecipazione di donne cittadine, espressione dell'utenza femminile, direttamente nei presidi pubblici e privati. Il coinvolgimento dell'opinione pubblica, in questo caso delle donne, per renderle nuovamente centrali e protagoniste attraverso l'espressione dei propri valori, delle proprie priorità e desideri, rappresenta, a nostro avviso, la chiave di volta di un'azione prolungata nel tempo, una vera e propria *road map* per abbattere questa epidemia, che è, al tempo stesso, sintomo e causa di sprechi e malasanità. Essa si consuma, ancora una volta, come crimine contro le donne e contro l'umanità dell'evento della nascita in nome di una medicalizzazione anestetizzante che tutto vorrebbe addormentare e manipolare, anche il desiderio di vivere, la forza di nascere e quella di partorire. nell'economia del dibattito, intervengo ora in discussione generale riassumendo anche la dichiarazione di voto per il Gruppo dell'UDC in questo contesto. La riflessione aperta con la discussione di differenti mozioni sulla cosiddetta medicina di genere rischia di essere, in maniera semplicistica, ridotta e rubricata ad argomento considerato troppo sensibile per colpire l'attenzione generale e, pertanto, fin troppo frettolosamente quanto facilmente ascrivibile al cosiddetto mondo delle rivendicazioni al femminile. Ma così non è. Il sostegno alla medicina di genere nasce dalla consapevolezza di quanto necessario sia rimuovere le varie forme di discriminazioni, più o meno evidenti, che impediscono la piena attuazione del diritto alla salute e ad avere, soprattutto, cure adeguate. dunque, di una semplice estensione di quote rosa alla sanità ma del riconoscimento più profondo, come rivelato dall'Organizzazione mondiale della sanità, dell'esistenza in campo sanitario di differenze di genere non tenute in debita considerazione e della necessità di adottare provvedimenti Sicuramente, l'Italia non è Paese in cui, per antonomasia, esistano eclatanti situazioni di palesi discriminazioni. Ma sarebbe sbagliato, comunque, non tenere conto dell'esistenza, nonostante ciò, di una molteplicità di fattori determinanti uno stato di sostanziale svantaggio delle donne in tema di tutela della salute. L'Organizzazione mondiale della sanità riconosce che dati biologici legati al sesso e dati di valenza socio-culturale legati al genere sono importanti e determinanti per la salute. Nella programmazione sanitaria nazionale emerge la mancanza di un approccio nuovo e complessivo ai temi della salute femminile. Occorre, pertanto, affrontare il problema con una diversa valutazione della programmazione e della produzione normativa sanitaria, capace di predisporre una risposta assistenziale più adeguata e che tenga conto dei molteplici fattori presenti. Non sono state, ad oggi, complessivamente affrontate e superate misconoscenze e sottovalutazioni. La scelta di temi scientifici, e persino di molte ricerche su malattie che colpiscono uomini e donne, ha di fatto ignorato le possibili differenze tra sessi. Se, infatti, le patologie strettamente femminili sono da anni al centro dell'attenzione dei gruppi di lavoro composti da donne, le cosiddette patologie miste, riguardanti cioè entrambi i sessi, richiamano la necessità di una valutazione di genere. Cancro, depressione, malattie cardiovascolari sono solo alcune delle patologie che colpiscono sia uomini che donne, ma non con la stessa modalità. Se è vero che nella interpretazione dei risultati si tiene conto della differenza tra maschi e femmine, è anche vero che, proprio nell'allestimento delle sperimentazioni cliniche si nasconde una differenza di genere difficilmente evidenziabile. Mentre all'uomo è attribuita una prevalenza di fattori ambientali, sociali e lavorativi tra le cause di malattia, alla donna è associata una prevalenza di fattori biologici e ormonali. Storicamente, quando erano messi a punto nuovi studi clinici, in particolare quelli relativi all'impiego di nuovi farmaci, erano coinvolti soggetti di sesso maschile. Ciò avveniva sia per la difficoltà nell'individuazione di un campione adeguato di donne negli studi clinici, sia per preoccupazioni relative ad interferenze indotte dalle variazioni ormonali, tipiche dell'organismo femminile, sull'effetto delle sostanze farmacologiche da testare, ma anche per la possibilità di esporre a rischi di tossicità donne potenzialmente fertili con conseguenti timori di procurare danni ai tessuti fetali. Per questa serie di motivi le donne in età fertile e le donne in gravidanza sono state sistematicamente escluse dalla maggior parte degli studi clinici. Pertanto, non avendo adeguatamente testato farmaci o presidi medico-chirurgici sulle donne, non esiste modo di conoscere quali siano state le reali condizioni di efficacia e di sicurezza sulle stesse. Ma è stato proprio questo doppio criterio di valutazione a penalizzare la donna. Sono sempre di più le evidenze scientifiche che rilevano differenze di comportamento e di risposta alle terapie in funzione del sesso, di cui si deve tener conto già nella messa in opera della stessa ricerca medica. Quindi, a fronte di una sempre maggiore esigenza di integrare in ogni pratica sanitaria il punto di vista di genere, la messa a punto di linee guida che integrino, nella sperimentazione farmacologica e nella ricerca medica, valutazioni relative ad entrambi i sessi, assume un'importanza fondamentale. Accanto al versante scientifico, l'altro ambito sul quale occorre concentrare l'attenzione resta sicuramente quello politico, in modo particolare parlamentare, dal quale emerge una grande attenzione al tema di provvedimenti legislativi più settoriali. Fino a pochi anni fa, le donne, nelle ricerche farmacologiche, venivano considerate dei «piccoli uomini», ritenendo quindi l'azione e l'utilizzo dei farmaci uguale nei due sessi, previo un semplice aggiustamento della posologia degli stessi. Non si è sentita l'esigenza di una sperimentazione riservata e dedicata alle stesse fino al 2002, cioè quando presso la Columbia University di New York è nato un settore specializzato nella medicina di genere.

nel corso della vita riproduttiva. A differenza di quanto sta accadendo in altri Paesi (come l'America e la Svizzera), in Italia, nell'ambito degli studi universitari, in particolare nella facoltà di medicina e chirurgia, non si è fatto ancora nulla per la costruzione di una medicina di genere, cioè di una medicina che tenga conto delle fisiologiche differenze, in modo tale da concretizzare tutti gli studi fin qui condotti sulla diversità del genere umano e raggiungere mete più precise ed incisive nella cura e nella prevenzione delle malattie. malattie. Non abbiamo alcuna intenzione di sostenere guerre di genere, perché sappiamo bene che il futuro appartiene ad altro piuttosto che a questo e che rispetto a tale profilo un'importanza fondamentale sta soprattutto nel riconoscere un ruolo alla genetica e alle biotecnologie. Nell'attesa, però, della predisposizione di una carta in cui possa essere scritto e riassunto il patrimonio genetico individuale, piuttosto che di genere, una carta che sia capace cioè di evidenziare, ad esempio, farmaci tollerati ma non altri, riteniamo giusto che questa Assemblea proprio ora, proprio all'inizio del suo mandato, si interroghi sul rilievo attribuito alla tutela della salute della donna e adotti ogni possibile iniziativa volta a superare le discriminazioni, le eccessive semplificazioni, le facilonerie e le storture della programmazione sanitaria. È per questo che sosteniamo le mozioni proposte.

sui problemi legati all'assistenza sanitaria e alla didattica dei corsi universitari e delle scuole di specializzazione. Le vostre mozioni intendono impegnare il Governo a istituire un corso di specializzazione in medicina di genere e chiedono il potenziamento delle misure predisposte per la tutela della salute delle donne. In relazione al primo profilo, le norme comunitarie e nazionali di settore prevedono la possibilità di istituire e attivare nuove scuole di specializzazione solo nei casi in cui dette scuole siano già presenti in due o o più Paesi dell'Unione Europea. In subordine, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 257 del 1991 dispone che possano essere attivati nuovi corsi di specializzazione solo per corrispondere ad obiettivi e specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda la fattispecie rappresentata dalle mozioni, si segnala che, secondo quando risulta al Ministero della salute, le Regioni non hanno ancora manifestato specifico interesse circa l'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina di genere. La procedura per l'istituzione e l'attivazione di una nuova scuola di specializzazione prevede il concerto tra i Ministeri della salute e dell'università e della ricerca, previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità. In ogni caso, le stesse mozioni rilevano che le problematiche relative alla specificità di genere femminile, intese come determinanti di salute, possono trovare, attesa la loro particolarità, adeguato riscontro esclusivamente tramite un approccio integrato che coinvolga trasversalmente tutti i settori delle scienze mediche, quali la ricerca, la pratica clinica, la diagnostica, la prevenzione. In considerazione di quanto sopra esposto, le citate questioni potrebbero trovare adeguate risposte tramite la revisione e l'adattamento ai nuovi scenari epidemiologici dei percorsi formativi e didattici del corso di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione medica, prevedendo al loro interno un'adeguata formazione sulla medicina di genere. Tale ipotesi permetterebbe sia di non disperdere il patrimonio di conoscenze sin qui acquisito, sia di ampliare e sviluppare gli studi e le ricerche attualmente in corso nelle materie di cui trattasi. Sarebbe così garantito un nucleo di conoscenze innovative che fungerebbero da volano per il trasferimento di queste nuove conoscenze e pratiche nel sistema della didattica, della formazione e dell'aggiornamento dei professionisti sanitari. Il Ministero della salute, peraltro, auspica che nell'ambito della specifica autonomia delle facoltà di medicina e chirurgia degli atenei italiani siano attivati corsi di aggiornamento e/o *master* universitari di medicina di genere. In relazione al secondo profilo, è da evidenziare che la tutela della salute della donna è un impegno di valenza strategica del Servizio sanitario nazionale, soprattutto in virtù del riflesso che gli interventi di promozione della salute, di cura e di riabilitazione in tale ambito hanno sul benessere psico-fisico nella popolazione generale, attuale e futura. Tale obiettivo è da sempre considerato prioritario nella programmazione sanitaria e ciò è ravvisabile sia nei vari Piani sanitari nazionali (di cui l'ultimo, relativo al triennio 2006-2008), sia nel progetto obiettivo materno - infantile, adottato con decreto ministeriale del 24 aprile 2000. L'azione del Ministero è ravvisabile in due azioni già avviate e in altre in corso Le prime, quelle già avviate, sono la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, cioè la legge finanziaria 2007, che ha istituito un fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale allo scopo di rimuovere gli squilibri sanitari tra le Regioni per il quale è stato stanziato un importo di 65,5 milioni di euro di cui 10 finalizzati ad iniziative per la salute della donna, iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato. Il Consiglio dei ministri ha approvato, inoltre, il 19 ottobre 2006, il disegno di legge recante norme in materia di tutela dei diritti della partoriente, promozione del parto fisiologico e salvaguardia sella salute del neonato che oggi è all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, dove si è concluso l'esame da parte del Comitato ristretto con l'elaborazione di un testo unificato.

L'obiettivo del progetto è definire e realizzare nel territorio nazionale un sistema di sorveglianza sui giovani in età evolutiva (sei-quindici anni) per acquisire in modo sistematico dati sui diversi stili di vita dei ragazzi, sui loro comportamenti in relazione ai principali fattori di rischio, in modo da realizzare una modalità di ascolto e di dialogo continuo, necessaria ad orientare gli interventi per la prevenzione e la promozione della salute e, più in generale, per costruire politiche giovanili strutturate sui loro reali bisogni. Per quanto concerne le azioni in fase di elaborazione sono da rammentare: la modifica del sistema di rilevazione dei dati statistici per genere e per indicatori socioeconomici; il piano per la promozione dello «Spazio Adolescenti» nei consultori familiari; il progetto «Apertura di sportelli contro la violenza sulle donne su tutto il territorio nazionale» all'interno dei pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza. È infine da ricordare che gli aspetti legati all'esigenza di tener presente la differenza di genere nell'organizzazione dei servizi sanitari, nella ricerca epidemiologica, nel trattamento delle patologie, come sottolineato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e la rilevanza, sotto il profilo sanitario e sociale, dei settori della prevenzione, della osservazione, della diagnostica, del trattamento e della riabilitazione, nonché dei fattori di rischio collegati ad alcune patologie emergenti tra la popolazione femminile, hanno costituito l'oggetto dei lavori delle varie commissioni dedicate da questo Ministero alla salute della donna. La più recente commissione istituita a tal riguardo ha terminato i propri lavori il 26 marzo 2006. È al momento in corso l'*iter* di costituzione della nuova «Commissione salute delle donne», che dovrà promuovere gruppi di lavoro specifici per definire, di concerto con le Regioni, le linee-guida per l'aggiornamento del POM e predisporre lo schema di piano nazionale triennale intersettoriale sulla salute delle donne. Tutte queste considerazioni servono, appunto, per

rompere questa specie di tabù, per cui sul pensiero delle donne, sulla socialità delle donne, sulle grandi questioni che le donne pongono, alla fine, intervengano sempre e solo le donne. Credo che il movimento femminista, l'autonomia della donna e le grandi innovazioni che hanno trovato posto nella società, nella cultura e nel pensiero - di cui parlerò dopo chiedono e interrogano anche gli uomini sul loro rapporto con la sessualità, con il potere, con gli altri sessi e sul loro rapporto con il mondo in genere.

sulla sua identificazione con il fallo e con le armi e quindi con il potere in quanto gestione delle vite altrui. Devo sottolineare che le donne, rispetto alla non neutralità del sapere, hanno insegnato a tutti che non esiste un'oggettiva verità, che non esiste una cosa che è di per sé valida comunque, ma che tutto deve essere relazionato nella quotidianità, negli affetti, nella vita, nelle esigenze

nella differenza, mantenendo sempre l'uguaglianza; infatti, la differenza è il solito trucco del potere per dividere e tenere le gradazioni del potere e della distribuzione della ricchezza

le soggettività che su questo si interrogano, senza la pretesa di avere risposte; ma già il fare le domande giuste in politica è una cosa enorme. Voglio concludere in positivo.

Contro le pulsioni di morte, contro le pulsioni distruttive ed autodistruttive, che sono parte dell'umanità e che non dobbiamo negare, dobbiamo mettere in campo la liberazione dell'amore, dell'amore grande, di eros, che vuol dire in questo caso l'aver cura, che è il più bell'augurio che si può fare ad una persona: abbi cura di te. Su questo il movimento delle donne e le donne, come pratica storica, hanno detto moltissimo.

un percorso che parta dalla propria soggettività, dalla differenza, dalla cognizione di quanto il potere maschile abbia perpetrato un'idea di potere, appunto, e di rapporti che ha sempre giocato sulla quantità e la negazione, da un lato, e sull'oppressione, dall'altro. Il movimento ecopacifista, con la sua grande idea del limite e della solidarietà, ed il movimento delle donne sono i due soggetti che pongono nuovi alfabeti di cui la prima parola è «empatia»: la capacità di sentire gli altri e di farsi carico delle pene, ma anche delle gioie, di tutti.

Forza Italia voterà a favore delle mozioni sulla medicina di genere, che mirano a colmare una grande carenza politico‑istituzionale relativa al tema della salute delle donne. Nella scorsa legislatura, in qualità di sottosegretario alla salute, ho aperto su questo tema (prima in Europa, lo dico con un certo orgoglio) un tavolo istituzionale che comprendeva l'Istituto superiore di sanità, l'AIFA, la cattedra di farmacologia, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari: l'ho fatto nella convinzione che fosse urgente avviare quelle ricerche necessarie per attuare una salute anche a misura di donna. Conoscere e riconoscere la diversità femminile significa migliorare la salute di tutta la popolazione. È tempo ormai che la politica, nella sua interazione con le società scientifiche, con l'industria farmaceutica, con gli operatori sanitari, con le associazioni dei cittadini, ponga fine ad un pregiudizio di genere dal punto di vista della ricerca e della salute pubblica. È tempo che cessi quell'errore metodologico in base al quale la maggioranza delle ricerche che sono destinate a comprendere la genesi e lo sviluppo delle malattie, che sono destinate a verificare la sicurezza e l'efficacia delle terapie, ignorava le donne e la loro biologica diversità. E non basta includere le donne negli studi clinici per utilizzare la terapia nel genere femminile, ma occorre studiare i farmaci anche in funzione delle variazioni ormonali che, come tali, possono influenzare la risposta alla malattia e ai farmaci stessi. Questa inaccettabile disattenzione non ha permesso - ed è questione assai grave - alle donne di avere la migliore terapia possibile. C'è poi da considerare che negli ultimi anni l'emancipazione delle donne e il diverso ritmo impresso nella loro vita ha portato una modifica sostanziale di alcune patologie che in passato colpivano maggiormente i maschi, ma che ora stanno diventando importanti cause patologiche e di morte per le donne. Si tratta in particolare delle patologie cardiovascolari e di alcuni tumori come quelli al polmone. Fino ad oggi, purtroppo, gli studi clinici più rilevanti che hanno portato alla registrazione di farmaci per tali patologie e la messa a punto di cure specifiche, sono stati disegnati e realizzati prevalentemente su soggetti maschili. Il riconoscimento delle differenze di genere è cosa recente nell'Organizzazione mondiale della sanità: il richiamo forte a questo tema da parte dell'OMS risale al 1998, per rilevare la complessa diversità dell'universo femminile anche in termini di salute e come questa diversità sia poco conosciuta e sostanzialmente sottovalutata. Il nostro Paese non può rimanere indifferente a quanto ci sia da fare per capire come il corso naturale delle malattie possa essere diverso tra i due generi, come l'uomo e la donna possano rispondere differentemente alle terapie e come la società possa rispondere in maniera diversa alla malattia della donna e dell'uomo. La Facoltà di medicina dell'università di Padova (la mia città) ha già iniziato un percorso molto importante, costituendo una commissione con implicazioni internazionali volta proprio ad approfondire questo tema. tema. Penso che il Governo non possa più perdere tempo per colmare il*deficit* di ricerca e di studi sulla salute delle donne, perché la pari opportunità

Signor Presidente, ringrazio i colleghi e le colleghe che hanno voluto restare in Aula per votare le mozioni Ci siamo trovati spesso in quest'Aula ad affrontare il tema della discriminazione femminile. L'abbiamo fatto però in altri ambiti e per altri argomenti. Oggi lo vogliamo fare rivolgendo una particolare attenzione al corpo e alle salute delle donne e vogliamo superare un bagaglio prezioso che ereditiamo dal passato. La donna nel rapporto con il corpo, con la propria sessualità e con sé stessa si è sempre occupata prima degli altri: il far stare bene gli altri, il portare e il donare la salute agli altri è stato l'obiettivo

La medicina ha sempre cercato di porsi, sia nella teoria che nella pratica, in maniera neutrale rispetto all'«essere uomo» o all'«essere donna», riconoscendo una specificità alle donne solo in relazione alla riproduzione. Questo ha provocato l'affermazione del principio dell'inferiorità biologica e naturale delle donne. Anche la ricerca medica ha orientato la sua attività verso il genere: tutta la metodologia, le argomentazioni, la raccolta e la successiva analisi dei dati focalizzano l'osservazione da un punto di vista maschile. Se una stessa malattia colpisce un uomo e una donna, l'uomo viene considerato il punto di vista privilegiato, la norma, il riferimento su cui formulare una valutazione dei sintomi, una prognosi e un'efficacia di trattamenti. In quest'ottica emerge un vizio di fondo che compromette gravemente la modalità di somministrazione delle cure offerte alle donne, proprio perché considerate differenti solo per quanto riguarda le capacità riproduttive. Questo pregiudizio della medicina, nei confronti della donna, viene definito, dagli addetti ai lavori, un "bias" di genere, un pregiudizio, appunto, evidente non solo nella scelta dei temi, ma anche nel disegno di molte ricerche. In medicina si parla per la prima volta della «questione femminile» nel 1991, quando l'allora direttrice dell'Istituto nazionale di salute pubblica americano, Bernardine Healy, pubblica due studi sul comportamento discriminante dei cardiologi nei confronti delle donne (credo che il Sottosegretario, che si occupa di cardiologia, conosca bene questo pezzo di storia). Le sue conclusioni evidenziavano una chiara discriminazione messa in atto dai cardiologi nei confronti del sesso debole. Nessuno pensò che la studiosa parlasse di discriminazione nel vero senso della parola, però i suoi studi portarono ad una riflessione nel mondo scientifico su quale valore

Lentamente la critica alla medicina, dal punto di vista di genere, si è spostata dalla cardiologia, fortunatamente, anche ad altri campi, come la psichiatria, la gastroenterologia, l'oncologia ed oggi, dopo non pochi anni, pochi anni, si comincia a parlare di approccio di genere e di medicina di genere. Le motivazioni dell'esclusione delle donne dalla ricerca scientifica, soprattutto quella relativa all'impiego di nuovi farmaci, hanno radici storiche: difficoltà nell'arruolamento e nel mantenimento delle donne negli studi clinici; preoccupazioni riguardo alle interferenze indotte dalle variazioni ormonali tipiche dell'organismo femminile sull'effetto delle sostanze farmacologiche da testare; da testare; preoccupazioni circa la possibilità di esporre a rischi di tossicità donne potenzialmente fertili, perché questo era l'unico destino sociale della donna; ma anche il timore di procurare danni a tessuti fatali. Tutte preoccupazioni giustissime; anzi, guai se non fossero preoccupazioni; ma non possono essere l'unico approccio. La necessità di testare un farmaco o un presidio medico-chirurgico direttamente sulle donne risulta evidente se si vogliono conoscere le reali condizioni di efficacia e di sicurezza su di loro. È essenziale ricordare che in medicina efficacia e sicurezza si misurano attraverso parametri fortemente correlati a variabili come l'età, il sesso, le caratteristiche di composizione dei tessuti, che a loro volta sono associati, in maniera specifica, alle caratteristiche biologiche legate al sesso, come gli ormoni, o alla prevalenza nei due sessi di particolari caratteristiche: corporatura, abitudini e stili di vita, concomitanza di disturbi più frequenti in uno dei due generi rispetto all'altro. La tutela e gli investimenti sulla salute della donna e sulla cura del suo corpo sono i tasselli fondamentali per la costruzione dell'uguaglianza di genere, ma anche per un significativo miglioramento delle condizioni di salute sia della donna

degli uomini e delle donne che operano in campo sanitario affinché la sua vita sia accompagnata dal benessere e dalla salute. La medicina però oggi non ha ancora ben chiara la prospettiva di genere e quindi non soddisfa al meglio i bisogni di salute delle donne e, indirettamente, nemmeno quelli degli uomini. Questo proprio a causa di un difetto di impostazione che difficilmente coniuga bene il confronto tra le necessità di salute dell'uomo e quelle della donna. Nel 2002, come hanno ricordato anche alcune colleghe, l'Organizzazione mondiale della sanità ha costituito il «Dipartimento per il genere e la salute della donna»,

socio-culturale - come fattori determinanti della salute. L'importanza di questo tema rende necessario un complesso di studi che possa operare per garantire un'uguaglianza nella medicina di genere e una corretta analisi delle differenze fisiologiche e culturali tra uomini e donne. In Italia, a livello universitario, nelle facoltà di medicina, non si è fatto nulla in questo senso e siamo ancora indietro rispetto agli Stati Uniti, dove la Columbia University di New York ha recentemente organizzato un corso specifico di medicina di genere, basato su un nuovo approccio che considera significanti le differenze biologiche tra uomini e donne. In Svizzera esiste un corso di laurea in medicina di genere presso la facoltà di medicina. La Comunità Europea, dal 1998, ha aperto un invito alle donne a partecipare ai programmi di ricerca e oggi esiste un settore della ricerca europea con un *focus* sulle donne. Nel 1999 è nato in Italia «Medicina Donna Salute», un gruppo di lavoro che ha dato un contributo importante al nostro Paese per l'individuazione e la comprensione della problematica di genere. Sempre in Italia, nel 2005 è nato

Quindi, ci sono tutti i presupposti affinché nel nostro Paese si ponga, con maggiore determinazione, l'attenzione su questo tema, perché non si può rimanere indifferenti davanti a questa assurda discriminazione di genere. Le pari opportunità possono realizzarsi solo in un'ottica di uguaglianza d'intenti, di analisi delle tipicità di genere nella tutela della salute e nel rispetto della persona umana. L'istituzione di un corso di studi specifico presso la facoltà di medicina

dell'Ulivo, che riteniamo utile e proficuo il dibattito di oggi e voteremo a favore di tutte le mozioni presentate perché, con sfumature ed angolature diverse, focalizzano, con attenzione ed intelligenza, il tema e consentono anche al Ministero

hanno sollevato alla Presidenza una questione relativa ai lavori di domani. Si chiedeva di sospendere

per vedere se era possibile posticipare la chiusura della seduta antimeridiana e quindi posticipare anche l'apertura e la chiusura della seduta pomeridiana di domani. I rappresentanti dei Gruppi presenti in Aula hanno assentito, salvo sentire i rispettivi Capigruppo, per cui si era pensato di chiudere la pomeridiana alle ore 17,30 e chiuderla alle ore 21. Ora, a prescindere dagli orari precisi, il senso era quello di recuperare un po' di tempo per consentire nel pomeriggio un inizio ritardato dei lavori. Vorrei chiedere alla Presidenza di verificare se questa disponibilità dei Gruppi permane, in modo che subito, anche domani mattina in apertura di seduta,

pomeridiana si aprirà alle ore 17 e si concluderà alle ore 21. Quindi, questa è la nuova scansione dei lavori del Senato di domani.

*(AN)*. Signor Presidente, colleghi, credo che non ci siano molti argomenti per illustrare la mozione, nel senso che essa non entra nel merito specifico di questo nuovo vaccino in grado di impedire l'infezione del papilloma virus. La mozione nasce da un'esigenza: considerato che tale vaccino è stato ritenuto necessario per

perché sicuramente è molto meno dispendiosa la prevenzione che non la cura, tenendo conto che ogni anno sono 550.000 i casi di cancro all'utero, cento dei quali al collo dell'utero, di cui responsabile è appunto questa infezione, con anche l'elemento drammatico di 1.700 vittime. Allora, se si vuole assumere un'iniziativa sociale di carattere preventivo e, e, paradossalmente, anche di risparmio economico, per il motivo che ho detto, credo che il Governo (ed è la ragione per la quale abbiamo proposto questa mozione) debba impegnarsi a far sì che tutte le giovani fino all'età compresa di 26 anni possano essere gratuitamente vaccinate. Signor Presidente, su circa 9 milioni di nuovi casi di cancro che ogni anno colpiscono la popolazione mondiale, il 18 per cento, vale a dire 1.600.000, sono causati da agenti infettivi. Il virus HPV è quello che causa il maggior numero di tumori: 550.000 l'anno; segue il batterio *helicobacter pilorii*, che è all'origine del cancro allo stomaco; ed il virus delle epatiti B e C, che possono causare il cancro del fegato. La ricerca scientifica spalanca le porte a nuovi orizzonti e offre speranze concrete di sconfiggere alcuni tipi di tumore che fino a pochi anni fa erano dei *big killer*, come il tumore al collo dell'utero. Questo tumore è la seconda causa di morte in Italia tra le giovani donne tra i 15 e i 44 anni, dopo il tumore al seno. Ogni anno, in Italia, muoiono circa 1.700 donne, cinque ogni giorno. Ogni anno i nuovi casi sono 3.500, cioè dieci casi al giorno. La Regione che fa registrare più casi è la Lombardia, seguono la Campania, il Lazio e la Sicilia. Nel 2003, si sono registrati 6.862 ricoveri per tumore maligno alla cervice uterina: un terzo di questi riguardavano giovani donne tra i 25 e i 44 anni ed un altro terzo le donne fra i 45 e i 64 anni.

essere colpite da questo tumore le penalizza fortemente. La Regione che ha fatto registrare il maggior numero di ricoveri è la Lombardia, seguita dal Lazio e dall'Emilia-Romagna. Quindi, l'annuncio della disponibilità di un vaccino per l'HPV è una grandissima notizia per tutte le donne. Le donne italiane conoscono il papilloma virus e il tumore del collo dell'utero. E ne hanno paura. Eppure non fanno prevenzione o perlomeno ne fanno molto poca. Le ragazze italiane tra i 25 e i 29 anni non si sottopongono al pap-test con regolarità, soprattutto al Sud. Più attente le donne tra i 45 e i 50 anni, in particolare le donne del Nord-Est. L'importanza di *screening* di massa e di qualità resta sempre l'arma vincente per arginare e curare tempestivamente questo tumore. Non è motivo di questa mozione, ma sulla prevenzione e sui piani di *screening* delle Regioni torneremo molto presto. Oggi ci occupiamo di vaccino. Con l'impegno della Commissione sanità il ministro Turco ha compiuto un importante passo nel campo della prevenzione, decidendo di vaccinare la coorte delle dodicenni. Già preannunciamo un emendamento alla prossima finanziaria per aumentare il finanziamento e ampliare il numero delle donne da vaccinare. Nel frattempo desideriamo occuparci di chi oggi, venuta a conoscenza di questa nuova scoperta, ma non appartenendo alla coorte delle dodicenni, desidera vaccinarsi. La casa produttrice vende il farmaco a 114 euro. A causa di quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, poi modificata con legge n. 289 del 2002, a tale costo viene aggiunto un rincaro del 6,65 per cento dovuto al grossista e del 26,7 per cento dovuto al farmacista. Costo finale in farmacia per una dose, 188,15 euro.

Quello che chiediamo a lei è di intraprendere ogni azione volta a contenere il costo finale di questo straordinario farmaco per quelle donne che non sono dodicenni e quindi si vogliono vaccinare, ma non appartengono alla corte delle dodicenni vaccinate sotto il Servizio sanitario nazionale.

predisporre azioni di sensibilizzazione delle donne in merito all'esigenza di una prevenzione per evitare di contrarre il cancro alla cervice uterina, nell'ambito del rafforzamento delle attuali campagne di informazione aventi ad oggetto i rischi connessi alle malattie infettive trasmissibili per via sessuale e le relative modalità di prevenzione, predisposte da pediatri di base, ambulatori pediatrici e consultori familiari.

«Oggi siamo qui per rinnovare il nostro impegno nell'informazione e nella diffusione capillare dei programmi di *screening*, ma anche per annunciare con soddisfazione che l'Italia sarà il primo Paese europeo a pianificare una strategia di vaccinazioni pubbliche contro il virus HPV e ciò avverrà contestualmente all'immissione in commercio nel nostro Paese di un nuovo vaccino contro il *virus* del papilloma umano che apre nuove prospettive per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina». Queste sono state le parole pronunciate presso la sala delle Conferenze del Senato dal ministro della salute Livia Turco qualche tempo fa, parole con le quali ha delineato l'impegno per la prevenzione del tumore della cervice uterina in occasione della presentazione della Campagna 2007 per la diagnosi precoce del tumore al collo dell'utero, promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. A seguito di ciò, l'Agenzia italiana del farmaco autorizzato in Italia, nel febbraio 2007, la commercializzazione del primo vaccino contro il papilloma virus (HPV). Il papilloma virus, malgrado possa essere prevenuto con una diagnosi precoce, determina il tumore alla cervice uterina e causa ogni anno, nel nostro Paese, 1000 morti tra le donne. La strategia di contrasto, basata sulla diagnosi precoce, da oggi aggiunge a tutto questo l'utilizzo di una attenta campagna di vaccinazioni mirate. La ricerca scientifica offre nuove frontiere: consente, attraverso le vaccinazioni, di prevenire anziché curare successivamente, e tutto questo implica anche una riduzione dei costi successivi per le cure. Le informazioni scientifiche oggi disponibili ci dicono che siamo in presenza di un vaccino sicuro, ben tollerato e in grado di prevenire, nella quasi totalità dei casi, l'insorgenza di un'infezione persistente dei due ceppi virali responsabili attualmente del 70 per cento dei casi di questo tumore. L'utilizzazione del vaccino rappresenta un importante presidio di prevenzione che si affianca, ma non sostituisce, lo *screening* periodico, attualmente raccomandato a donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni. II vaccino attuale risulta attivo contro il 70 per cento dei virus associati al carcinoma uterino, ma per il restante 30 per cento permane ancora, come unica prevenzione, il pap-test. Esistono in diverse Regioni italiane programmi di *screening* gratuito effettuati ogni tre anni e rivolti a tutte le donne di età compresa fra 25 e 64 Gli studi realizzati fino ad oggi hanno coinvolto donne di età inferiore a 26 anni che non erano state contagiate dal virus, e per le quali si è evidenziato che la vaccinazione risulta efficace nel prevenire il 98 per cento dei casi di infezione. Il vaccino, che ha lo scopo di prevenire l'infezione, ma non di curarla, a seguito della disposizione del Ministero della salute, è previsto che venga gratuitamente offerto, così come ricordato precedentemente, a tutte le bambine di 12 anni di età. prevede un'iniezione intramuscolare, ma di questa ne sono previste 3 dosi: la seconda dopo 2 mesi e la terza dopo 6 mesi dalla prima. Ora, va evidenziato che, nonostante il notevole passo in avanti compiuto, emerge ancora forte la preoccupazione che, essendo esentate dal costo d'acquisto soltanto le dodicenni, l'elevato prezzo finale del vaccino, pari a 188,15 euro a dose (moltiplicato per tre dosi in un anno), possa comprometterne e ridurne l'acquisto. Pertanto, sembra doveroso e necessario, pur nella consapevolezza che la vaccinazione rappresenta un alleato importante ma non esclusivo per ridurre il rischio di tumore, che il Governo faccia fino in fondo la sua parte ed intraprenda ogni azione utile per promuovere quanto più possibile la diffusione e l'acquisto del vaccino, al fine di abbattere il costo del prodotto anche per tutte le donne e adolescenti di età compresa tra i 13 e i 26 anni. Evidentemente, a seguito di quanto esposto, il Gruppo UDC voterà a favore della mozione proposta.

ministro della salute Livia Turco ha adottato un programma di vaccinazione non obbligatoria limitato alle ragazze di 12 anni di età perché questo, da studi di evidenza clinica, è il momento giusto. Infatti, si tratta innanzitutto di un vaccino precauzionale, senza efficacia se somministrato a una donna che abbia già contratto il *virus*.

Bisogna sapere che il vaccino non dà una copertura totale dal rischio di contrazione del papilloma virus e, quindi, dai rischi connessi di contrazione di un carcinoma a seguito dell'infezione da papilloma virus. Ritengo che questo vada detto e che quindi non sia solo un problema di aumento generalizzato delle coorti di donne che si sottopongono alla vaccinazione né di aumento dell'età. Credo che esista un problema di informazione corretta, e anche di sensibilizzazione, soprattutto sui rischi connessi a tutte le malattie infettive trasmissibili per via sessuale e sulle relative modalità di prevenzione, compreso, per l'appunto, il pap-test e lo *screening* triennalmente suggerito. Questo perché non si creino aspettative illusorie, che potrebbero generare, nel tempo, Dobbiamo poi affrontare il tema del monitoraggio dell'efficacia nel tempo del vaccino e, soprattutto, verificare cosa succederà, in somministrazione del vaccino, dei ceppi non colpiti dallo stesso, che potrebbero diventare più resistenti. Dunque, deve esser chiaro che il vaccino è efficace se somministrato nelle idonee condizioni di tempo e di luogo e, soprattutto, in un contesto di corretta informazione. la copertura totale dal rischio e, poiché il nostro obiettivo è di ridurre il rischio anche per quel 30 per cento di casi che non è coperto dal vaccino, riteniamo che esso debba essere somministrato,

integrando quanto ha avuto modo di esporre il primo firmatario della mozione, senatore Tofani, e anche alla luce delle considerazioni di altri colleghi, questa sera è importante discutere di un tema che riguarda migliaia di persone. Basta solo immaginare che, ogni anno, in Italia, sono diagnosticate 47.000 lesioni di basso grado al collo dell'utero, pari a 130 casi al giorno, e che, come diceva il collega Tofani, sono 14.700

ha annunciato che l'Italia sarebbe stato il primo Paese ad approvare il vaccino contro il papilloma virus umano e, contemporaneamente, a raccomandare la vaccinazione gratuita di tutte le dodicenni a livello regionale. Il 3 marzo, l'Agenzia italiana del farmaco pubblica il decreto con cui si pone in commercio il vaccino, che infatti è disponibile nelle farmacie italiane dal 28 marzo 2007.

intanto, e ci auguriamo che il sottosegretario Gaglione ci risponda, cosa è stato fatto per agevolare le Regioni ad avviare le campagne di vaccinazione contro il papilloma virus umano per le dodicenni e quando partiranno le campagne di vaccinazione a livello regionale. So che

il Consiglio superiore, l'ulteriore sviluppo della strategia vaccinale dovrebbe prevedere un'evoluzione modulare con estensione ad una seconda coorte di donne di 25-26 anni di età,

Il primo vaccino per la prevenzione delle lesioni precancerose del carcinoma della cervice, delle lesioni displastiche della vulva e dei condilomi genitali è stato recentemente autorizzato con procedura centralizzata europea. Con determinazione del 28 febbraio 2007, l'Agenzia italiana del farmaco ha deliberato sul regime di rimborsabilità e sul prezzo di vendita del vaccino anti-HPV Gardasil. Il vaccino è stato classificato in classe HRR, cioè a dispensazione attraverso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, medicinale soggetto a prescrizione medica. è prevista la gratuità per le bambine nel corso del dodicesimo anno di vita ed è sottoposto a sorveglianza e monitoraggio da parte dell'Istituto superiore di sanità. Si precisa, inoltre, che presso l'Agenzia europea dei medicinali è in corso la valutazione di un vaccino bivalente contro l'HPV 16 e 18. L'infezione da HPV è la più comune tra le malattie sessualmente trasmesse. Si stima, infatti, che oltre il 75 per cento delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della vita con un virus HPV e il 50 per cento delle donne si infetti con un tipo a rischio oncogeno. Tuttavia, la maggior parte delle infezioni è transitoria, perché il virus viene eliminato dal sistema immunitario, prima di sviluppare un effetto patogeno. In caso di infezioni persistenti, la progressione verso le lesioni precancerose e il tumore richiede comunque molti anni. In particolare, l'intervallo tra le lesioni precancerose iniziali della cervice uterina e l'insorgenza del carcinoma può essere di decenni. Lo *screening* per il carcinoma della cervice, consente quindi di identificare le lesioni precancerose e di intervenire prima che evolvano in carcinoma, il più comune pap-test. Infatti, nelle nazioni che hanno avviato i programmi di *screening* organizzati, basati sull'offerta del pap-test, si è assistito, nelle ultime decadi, ad un importante decremento dell'incidenza di queste neoplasie. Attualmente, nel nostro Paese, la prevenzione del carcinoma è basata esclusivamente sul pap-test, raccomandato ogni tre anni per le donne tra i 25 e i 64 anni. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale *screening*, l'adesione ai programmi organizzati di *screening* della cervice è andata aumentando nel tempo. L'infezione da HPV viene acquisita abbastanza precocemente, nel corso dei primi anni di attività sessuale. Pertanto, il modo più razionale ed efficiente di impiegare questo nuovo vaccino è quello di offrirlo attivamente subito prima dell'inizio dell'attività sessuale, inducendo così una protezione elevata prima di un eventuale contagio da HPV. Tale scelta strategica, d'altronde, è coerente con i principi della prevenzione vaccinale, il cui successo si fonda proprio sulla protezione immunitaria prima dell'esposizione all'agente infettivo. Considerando le evidenze scientifiche attualmente disponibili e coerentemente con le raccomandazioni della Organizzazione mondiale della sanità, contestualizzate nella realtà italiana, il dodicesimo anno di vita risulta il più indicato per effettuare la vaccinazione, in quanto il beneficio è massimo proprio nelle preadolescenti. In questa fascia di età, infatti, è stata osservata la migliore risposta immunitaria al vaccino e la probabilità di aver contratto l'infezione è molto bassa poiché, nella maggior parte dei casi, non ha avuto ancora inizio l'attività sessuale. tenuto conto che la vaccinazione è controindicata in gravidanza, evento raro a questa età, non sono necessarie precauzioni per evitare che insorga una gravidanza nel corso dei sette mesi necessari al completamento del ciclo vaccinale. Non si deve infatti dimenticare che, affinché il vaccino garantisca una protezione efficace, è necessario che il ciclo a tre dosi previsto venga rispettato e completato. Ancora, all'età di 11 e 12 anni, in concomitanza con la scuola dell'obbligo, è più facilmente realizzabile l'offerta attiva. Viceversa, i tassi di copertura si riducono inevitabilmente nelle fasce d'età successive, e, così come per le altre vaccinazioni, è da attendersi che la mancata vaccinazione si concentri nelle classi sociali più svantaggiate, che sono a maggior rischio sia di sviluppare l'infezione, sia di un mancato ricorso allo *screening*. Non si può trascurare, inoltre, un importante aspetto organizzativo: l'offerta delle vaccinazioni in questa fascia d'età comporta che essa venga praticata presso quegli stessi servizi già impegnati nelle vaccinazioni per l'infanzia, mantenendola nell'ambito del patrimonio professionale e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, anche a garanzia di equità, di accesso alla prevenzione vaccinale per la popolazione *target*. Inoltre, l'offerta vaccinale all'età di 12 anni può essere ottimizzata sfruttando l'occasione del richiamo previsto, tra 11 e 15 anni per la vaccinazione antidifterica e antitetanica, o in occasione del recupero della seconda dose del vaccino antimorbillo, parotite e rosolia. Le possibili strategie sono state recentemente discusse anche dal Consiglio superiore di sanità, che ha espresso all'unanimità il parere che la vaccinazione delle ragazze nel dodicesimo anno di età rappresenti, per il contesto italiano, la migliore strategia vaccinale. Con decreto del Capo del Dipartimento della prevenzione e comunicazione del Ministero della salute del 27 febbraio 2007, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di raccomandazioni nazionali per la vaccinazione anti-HPV. Il gruppo, nel quale sono presenti i rappresentanti dell'AITA e dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni, delle società scientifiche e delle categorie professionali tradizionalmente impegnate nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie croniche o degenerative dell'apparato riproduttivo femminile, ha mandato di predisporre una strategia vaccinale e definire precisi indirizzi ai servizi e agli operatori per garantire equità d'accesso e parità di offerta attiva a tutta la popolazione *target* su scala nazionale. Il gruppo, tenuto conto anche del parere tecnico-scientifico espresso dal Consiglio superiore di sanità, ha predisposto il documento «Proposta di strategia per l'offerta attiva del vaccino contro l'infezione da HPV in Italia».